La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario fino al 5 luglio. Oggi pomeriggio proseguirà il dibattito e avranno luogo le votazioni sulle mozioni e gli ordini del giorno concernenti gli studi di settore. Se possibile, se ce ne sarà il tempo, riprenderanno inoltre le votazioni sul disegno di legge recante delega in materia di sicurezza sul lavoro.

28 giugno sarà discussa e votata la mozione Salvi ed altri sulla Conferenza internazionale sul sistema giudiziario afgano. Potrà intervenire un oratore per Gruppo. Dopo il voto della mozione, sempre giovedì mattina, sarà avviata la discussione generale del disegno di legge in materia fiscale con il voto delle eventuali questioni incidentali. La discussione generale proseguirà poi - fino alla sua conclusione - giovedì pomeriggio. Per quanto riguarda la prossima settimana, i lavori riprenderanno a partire dalle ore 10,30 di martedì 3 luglio con l'inizio della discussione generale della legge comunitaria, fino alla fine della seduta antimeridiana. Nel pomeriggio proseguirà la discussione del disegno di legge in materia fiscale, auspicabilmente fino alla sua conclusione. Mercoledì 4 luglio, dalle ore 9,30 alle ore 10,30, nell'Aula del Senato avrà luogo, alla presenza del Capo dello Stato, la commemorazione di Giuseppe Garibaldi in occasione del duecentesimo anniversario della nascita. La seduta avrà pertanto inizio alle ore 10,30 con l'avvio della discussione generale del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario che proseguirà per il resto della settimana, incluso il pomeriggio di giovedì 5 luglio, ad eccezione delle seguenti "finestre": a fine seduta antimeridiana di mercoledì 4 saranno poste ai voti le dimissioni presentate dai senatori Vernetti, Magnolfi e Selva; giovedì 5, dalle ore 9,30 alle ore 11,30, sarà esaminato il disegno di legge sulla nomina elettiva dei giudici di pace, fatto proprio dal Gruppo della Lega in quota provvedimenti delle opposizioni; alle ore 20,30 interpellanze e interrogazioni. Avverto infine che domani, alle ore 12,15, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale, quinto scrutinio a maggioranza dei tre quinti dei componenti. Voteranno per primi i deputati; la chiama dei senatori inizierà intorno alle ore 13,45.

Ecco, mercoledì c'è questo grosso avvenimento a Torino della dichiarazione del sindaco Veltroni. Le confesso, Presidente, che noi vorremmo esserci per poter ascoltare in diretta; mi sembra che ci siano tanti altri personaggi. Le chiediamo veramente, proprio per diminuire questa tensione che sentiamo dentro, di darci la possibilità di partecipare,

Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, onorevole sottosegretario Lettieri, ci troviamo qui, a distanza di sole tre settimane dall'ultimo appuntamento (mi riferisco all'*affaire* "generale Speciale-Guardia di finanza") per discutere l'ennesimo fallimento della premiata ditta Prodi-Visco sul piano della politica fiscale, a dare voce alla protesta degli artigiani e del popolo delle partite IVA, che, soprattutto nelle parti economicamente più vivaci del Paese, nelle ultime settimane si stanno ribellando alle modifiche agli studi di settore che avete apportato con l'ultima finanziaria. Dobbiamo ricordare innanzitutto che gli studi di settore sono stati introdotti nel nostro ordinamento con la finalità di far emergere il sommerso attraverso un rapporto di fiducia e collaborazione tra contribuente, associazioni di categoria e amministrazione finanziaria dello Stato, vista non più come esattore Moloch, ma come una parte dello Stato della quale si può cominciare ad avere fiducia e con la quale si può finalmente dialogare. E' sempre stata questa la filosofia in materia fiscale che sotto la sapiente regia del ministro Tremonti ha ispirato l'azione del Governo Berlusconi; condoni sì, ma anche riduzione delle aliquote, aumento della *no tax area*, eliminazione di tasse inutili, snellimento e semplificazione delle procedure, applicazione dell'accertamento per adesione, rispetto dei diritti del contribuente. E i risultati si sono visti, con la progressiva emersione di un sommerso, che in precedenza sfuggiva, da cui è derivato un extragettito per l'esercizio 2006. Questo approccio, come dire, di leale collaborazione fra contribuente e Stato, che ha ispirato tutti i cinque anni del Governo Berlusconi, è stato da voi gettato alle ortiche alla prima occasione: la finanziaria per il 2007! Presi dall'ansia giustizialista del vice ministro Visco, animati come siete dall'odio di classe e all'insegna dell'ormai famoso *slogan* di Rifondazione Comunista, che ha tappezzato i muri del Paese, con un bel panfilo in primo piano, che recitava «perché anche i ricchi piangano», intendendo ovviamente per ricchi tutti coloro che denunciano un reddito superiore ai 40.000 euro lordi l'anno, avete violato tutti i patti sottoscritti con i contribuenti, innalzato immotivatamente le aliquote fiscali e fissato unilateralmente nuovi indicatori di normalità economica, senza alcuna concertazione con le associazioni di categoria delle piccole e medie imprese e degli artigiani. E' stato infatti aggiunto, ai concetti di congruità e di coerenza, appunto l'indice di normalità, ovvero di vicinanza ad una teorica ed astrusa media statistica frutto di improbabili regressioni matematiche e di proiezioni virtuali. Ma la cosa più grave è che questi parametri sono stati applicati con effetto retroattivo ai redditi del 2006, in dispregio all'elementare principio di irretroattività delle norme fiscali, principio sancito peraltro anche dallo Statuto del contribuente. I risultati dell'applicazione di questi nuovi parametri determinano conseguenze assurde e vessatorie, ma soprattutto collidono con il buon senso e la logica ed hanno determinato una rabbia dei contribuenti. Prima di pronunciare questo intervento, sottosegretario Lettieri, ho voluto documentarmi in modo scrupoloso e ho portato con me una documentazione che sono pronto a mettere a disposizione del Governo, ove ritenesse di contestarla. Allora, sottosegretario Lettieri, mi dica se è mai possibile, e oserei dire giusto, che il titolare di un'attività di installazione di impianti idraulici di Vicenza, che nel 2005 era congruo con euro 223.000 di ricavi e che nello stesso anno dichiarava ricavi per euro 249.000, ora con l'applicazione dell'indicatore durata delle scorte dovrebbe esporre per l'anno 2006 maggiori ricavi per oltre 67.000 euro. Uno strabiliante 30 per cento in più che appare privo di qualsivoglia logica e ragionevolezza! Quale giusta causa motiverebbe mai, a suo giudizio, un adeguamento così sensibile? Forse gli indicatori economici dell'ultimo anno giustificano un aumento così drastico? O a giustificare tale adeguamento è solo la *vis* punitiva del vice ministro Visco, ormai il più impopolare fra gli esponenti del Governo in carica, come certificano i più recenti sondaggi? Ma posso documentare anche altre situazioni ancora più assurde. Per il titolare di un'attività di rivestimento di pavimenti assolutamente marginale, sempre di Vicenza, con ricavi dichiarati nell'anno 2005 per euro 13.296, lo studio di settore prevede addirittura un adeguamento del dichiarato pari al 110 Se ritiene potrei continuare con altri esempi pratici; come le ho detto prima, sono molto documentato. Sono queste le cause della rivolta fiscale che si è accesa nel Paese e soprattutto al Nord! È mai possibile che con questi indici circa il 60 per cento delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi nel 2006 rischiano di risultare non congrui? È mai possibile che le aziende che realizzano investimenti, quelle di recente costituzione e quelle che fanno ricerca (che quindi si dovrebbero considerare meritevoli di particolare sostegno), siano praticamente tutte fuori dai parametri che avete introdotto? Non vi viene il dubbio di aver partorito un mostro? Siete consapevoli del disastro che avete combinato? Signor Sottosegretario, condividiamo tutti l'esigenza di combattere l'evasione fiscale, ma non è certo la faccia truce e vessatoria del fisco, che si manifesta nel corso degli accertamenti della Guardia

nel corso di una recente audizione presso la Commissione finanze della Camera, ha avuto l'ardire di affermare che chi non si adegua agli studi di settore alla fine dell'accertamento paga il triplo di quanto avrebbe fatto di quanto avrebbe fatto aderendo spontaneamente. Se manterrete le aliquote fiscali agli attuali livelli confiscatori, che non trovano paragoni nelle economie avanzate; se, come si dice, volete addirittura innalzare a breve il prelievo fiscale sui titoli di Stato, le conseguenze saranno disastrose per il sistema Paese. L'evasione fiscale sarà sempre più percepita da una larga fetta di contribuenti come l'unica difesa da un fisco ingiusto e vessatorio. Lo sciopero fiscale di intere aree del Paese è una prospettiva che deve allarmare tutti, ma è un rischio concreto se ragionevolezza e buon senso non prevarranno. Con la strada che avete deciso di percorrere, con la lotta di classe, alimentando l'odio sociale, l'unico risultato che otterrete è quello di costringere le aziende marginali a chiudere, a ritirarsi nel sommerso, ed in generale a frustrare investimenti, emersione e crescita dimensionale delle aziende. Gli studi di settore che avete predisposto costituiscono soltanto uno sfregio alla civiltà del diritto, nel momento in cui pretendete, loro tramite, di predeterminare unilateralmente e automaticamente l'ammontare dei ricavi da dichiarare, sulla base non del reddito effettivo, ma del reddito presunto del contribuente. Per questo con la mozione oggi all'esame del Senato chiediamo al Governo di sospendere per l'anno in corso l'efficacia di tali strumenti, di eliminare l'odiosa retroattività delle norme e di aprire immediatamente un tavolo concertativo con le associazioni di categoria del lavoro autonomo, degli artigiani, delle piccole e medie imprese. A conclusione del mio intervento, mi rivolgo, signor Presidente, in particolare a quei parlamentari dell'altro schieramento che di questa battaglia hanno dichiarato di condividere molti punti. Mi riferisco, ad esempio, alla senatrice Rubinato, che pure è veneta e proviene dalla Provincia di Treviso, particolarmente sensibile a questi temi, la quale, con alcune prese di posizione, ha conquistato di recente ampi spazi sul più diffuso quotidiano economico nazionale; alla stessa collega senatrice Thaler Ausserhofer, che ha portato avanti nelle ultime settimane una coraggiosa battaglia personale per un fisco più giusto; al senatore Pinzger, di cui ho apprezzato l'intervento stamane, e a tanti altri moderati del centro-sinistra che sappiamo condividono le nostre preoccupazioni. Ebbene, colleghi, abbiate il coraggio di lasciare da parte le logiche di schieramento e oggi contribuite con noi a convincere il Governo a modificare una politica fiscale che riconoscete sbagliata e vessatoria. I nostri elettori ci osservano, attendono da noi coerenza di comportamenti e magari in questa occasione un lavoro comune. *(Applausi

debbo dire a tradimento, della logica degli studi di settore; il secondo è il contesto di politica fiscale ed economica nel quale questo provvedimento si colloca.

applicate retroattivamente, determinano che soggetti che avevano dichiarato un reddito che rispettava i parametri che lo Stato aveva loro indicato nel raccordo e nel rapporto tra fisco e contribuente e che quindi erano dichiarati dallo Stato

*ex post*, tre milioni e mezzo di contribuenti italiani che l'anno scorso avevano rispettato le regole con il decreto di marzo si Ciò implica una gigantesca ipocrisia da parte del Governo e di tutti noi che rappresentiamo i cittadini e gli elettori in Parlamento, per la banale considerazione che tre milioni e mezzo di soggetti che, secondo le precedenti norme, erano in regola, nel momento in cui hanno scritto i numeri del loro reddito e del loro bilancio si trovano fuori regola e sono soggetti ad accertamento. Cari colleghi, il nostro sistema dell'Aministrazione finanziaria, se lavora a pieno ritmo tutto l'anno, determina una capacità di accertamento che, nella migliore delle ipotesi, arriva a 100.000 soggetti. Questa è la grande ipocrisia. Come si può pensare di sottoporre ad accertamento tre milioni e mezzo di soggetti, a fronte di una capacità amministrativa di 100.000 accertamenti? Significa che, al che, al ritmo di 100.000 soggetti all'anno, dovremmo continuare ad accertare i redditi del 2006 Ma ci rendiamo conto della stupidaggine e della ipocrisia che vengono a determinarsi? Vi chiedo di essere seri, perché se caso mai i normali cittadini capissero questi banalissimi dati, avrebbero motivo non per una rivolta fiscale, ma per una rivolta verso le istituzioni democratiche del Paese. Questo è ciò che sta avvenendo e nessuno dice nulla. D'altra parte, nella stessa finanziaria la vessazione verso i piccoli operatori

Nello stesso vostro provvedimento agevolate le poche (tre o quattro) grandi società di intermediazione immobiliare e sottoponete a vessazione, definendoli evasori, coloro che, in base alle regole, erano in linea con il fisco, e lo fate *ex post*. Non siamo al primo caso, perché è nella logica della sinistra, di questa strana sinistra italiana, connivente con i grandi gruppi, con le grandi banche e con la grande finanza nazionale ed europea. Non è la prima volta. Basti ricordare che nella vostra legislatura 1996-2001 il ministro Visco introdusse l'IRAP per le piccole e medie imprese, la DIT e la superDIT per i grandi gruppi;

e ben più approfonditi elementi di giudizio. Per questo la mozione n. 110 (testo 2) è un atto dovuto del Parlamento, non dell'opposizione: è nell'interesse vostro di maggioranza non andare a raccontare ai cittadini balle ed ipocrisie. Non vi lamentate se poi i cittadini italiani, che non sono tutti fessi, si accorgono e vi tolgono il consenso; per quello che ci riguarda, il consenso che avete perduto ad oggi già basta ed avanza. secondo luogo, signor Presidente, mi appello a lei, al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte dei conti, lo faccio formalmente in un'Aula del Parlamento, dopo averlo fatto più volte in quest'Aula, più volte anche usando usando la comunicazione di massa. Questo provvedimento si innesta in un contesto, il che non era mai avvenuto nella storia della Repubblica italiana, italiana, di totale incertezza e approssimazione delle risultanze contabili del bilancio dello Stato e del quadro della finanza pubblica italiana. È ora di finirla. È cominciato tutto con il precedente DPEF, quando il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'economia ci raccontarono che i conti erano allo sbando; a settembre fu presentata la relazione previsionale e programmatica e la proposta di disegno di legge finanziaria; a settembre il Governo ha scritto

che le spese complessive per il 2007 sarebbero state 746 miliardi di euro e che il *deficit* pubblico sarebbe stato del Presidente, faccio riferimento a documenti ufficiali, non come affermò in quest'Aula il ministro Padoa-Schioppa, in risposta a queste mie stesse considerazioni a dicembre, dicendo che erano fantasie del senatore Baldassarri: sono riscontri contabili del Governo. A dicembre sostenemmo e continuo a sostenere che viviamo - ormai da sei mesi - con un bilancio dello Stato falso sul fronte delle entrate e sul fronte delle spese; non falso perché è una mia personale valutazione, ma sulla base dei riscontri contabili resi disponibili dal Governo. Dissi a dicembre che, sulla base dei calcoli del Governo, lo stesso avrebbe dovuto scrivere per il 2007 un gettito complessivo di 726 miliardi, di 23 miliardi superiore a quello che ancora oggi è scritto nel bilancio pubblico, cioè 703 miliardi Il Governo si rifiutò; ci spieghi allora perché otto settimane dopo, senza nessun ulteriore riscontro contabile del 2007, il Governo scopre all'improvviso che il gettito 2007 non è più di 703 ma di 713 miliardi - e lo scrive

il Governo è impegnato a presentare il bilancio di assestamento in corso d'anno: è l'ultimo atto formale obbligatorio possibile per sanare il *vulnus* di avere un bilancio dello Stato Mi rendo conto delle preoccupazioni del ministro Padoa-Schioppa, perché ovviamente il «tesoretto», così come lui lo definisce, o il «falso in bilancio», così come la regola contabile imporrebbe di chiamarlo, a tutt'oggi non è incorporato nel bilancio dello Stato: alle ore 17 del 26 giugno troviamo ancora scritta la

Capisco le preoccupazioni di Padoa-Schioppa, perché lui per primo sa che con la legge finanziaria ha nascosto le entrate, ma ha anche determinato 35 miliardi in più di spesa pubblica corrente. Ilministro Padoa-Schioppa sa che in questi giorni, per tenere in piedi per qualche settimana in più questo Governo e questa maggioranza, sta determinando un ulteriore sbracamento di 9-10 miliardi di aumento della spesa corrente. il Ministro dell'economia, che sta facendo un ulteriore imbroglio, non solo sui conti, ma anche verso i lavoratori, perché quando viene a profilarsi, per la riforma delle pensioni, un accordo sinistra cosiddetta alternativa e antagonista, connivente con questo imbroglio ai lavoratori, se dovesse emergere un accordo a quota 96,

e quindi andrebbe in pensione dopo due o tre anni. È un altro trucco, altro fumo che state buttando sugli occhi dei lavoratori, e mi meraviglio ancora che la cosiddetta sinistra antagonista, che nel programma dell'Ulivo aveva fatto scrivere: «Eliminazione dello scalone», punto, possa ancora una volta accosciarsi pur di rimanere attaccata a quella posizione. A tutto questo aggiungo un dubbio: quanto costerà questo passaggio in termini di ulteriori fondi all'Alto Adige? Abbiamo vissuto in quest'Aula un fatto scandaloso: mentre un rappresentante di quel Gruppo attaccava il Governo su tutti i fronti ad alzo zero, un altro rappresentante contrattava sui banchi del Governo quanti soldi per comprare quei voti! Abbiamo vissuto in prima persona questo, dentro un'Aula parlamentare. Signor Presidente, questo è il contesto, questi sono provvedimenti. Mi appello a lei, mi appello ancora al Presidente della Repubblica perché è la massima magistratura dello Stato, mi appello al Presidente della Corte dei conti perché è la massima magistratura contabile: è ora di smetterla con questo balletto! Cifre che appaiono la mattina non ci sono il pomeriggio, articoli di giornale con i quali si allude ad un «rischio manovra» da 8-10 miliardi e il ministro dell'economia, addirittura lancia l'allarme «conti pubblici» e stiamo discutendo in una condizione nella quale sfido ogni collega del Senato, ogni collega della Camera e molti Ministri a farci sapere se ciascuno di loro è in grado di conoscere non dico il dettaglio del bilancio pubblico, ma le grandi cifre, quanto è il totale delle entrate, quanto è il totale delle spese, quanto è il totale del *deficit*. Si profila addirittura, adesso, la possibilità di chiudere il 2007 con un *deficit* ancora più basso di quanto era stato previsto, perché i conti dicono che potremmo attestarci la legge finanziaria che, al comma 4, stabilisce che ogni eventuale maggior gettito deve andare a ridurre il *deficit* e il debito. E sento dire sento dire - purtroppo dobbiamo seguire i giornali, perché il Governo in quest'Aula non ha mai dato le informazioni, ma le fa trapelare dai giornali - che si potrebbe ritoccare il *deficit* di quest'anno da 2,1 a 2,5 (cosa vuoi che sia uno 0,4 in più?) per chiudere la baracca, il mercato, il *suk* politico che si sta svolgendo ancora una volta in questi giorni fuori da quest'Aula, magari all'insaputa della stragrande maggioranza degli stessi senatori della maggioranza. Questo *suk* deve finire: la certezza dello Stato di diritto poggia anche sulla certezza del bilancio dello Stato e dei conti pubblici. Siamo a giugno e non sappiamo ancora qual è la cifra da scrivere in bilancio. Io aspetto il bilancio d'assestamento, non il DPEF, perché che senso ha discutere un DPEF se non c'è la pietra d'appoggio che sono i conti del 2007? Poi penseremo al 2008, al 2009 e al 2010, ma se i conti del 2007 ad oggi sono talmente ballerini, come credo di aver già ampiamente dimostrato, ebbene, il Governo abbia un sussulto di dignità, di senso istituzionale: ci porti un bilancio d'assestamento con le cifre vere, con i numeri veri, e su quella base si potrà discutere, eventualmente, il DPEF. Se così non fosse, ci assumeremmo tutti una responsabilità storica, istituzionale, di aver fatto passare l'intero anno 2007 con il bilancio pubblico falso sulle entrate, falso sulle spese e falso sul *deficit* pubblico. Infatti, cari colleghi, può significare poco qualche decimale, ma se casomai chiudessimo il 2007 con il 2,5 per cento

alla fine della precedente legislatura il *deficit* ben al di sotto del 3 per cento, si inverte la tendenza e subito, al primo anno della nuova legislatura, il *deficit* pubblico sarebbe nel 2007 più alto che nel 2006. Questo significa che basterebbero 50 punti base, cioè lo 0,5 per cento, di effetto automatico sull'andamento dei tassi d'interesse relativi ai titoli di Stato italiani, per avere con un debito pubblico al 107 per cento, tra i 12 e i 13 miliardi di oneri per interessi in più. quindi penalizzato le nuove generazioni, non sostenuto le generazioni correnti, e rinviato il problema al futuro, a quelle nuove generazioni alle quali stiamo dicendo che chi va in pensione adesso va in pensione con il vecchio sistema di partizione e a regime all'80 per cento di retribuzione,

pensionabile oggi significa chiedere a chi sta per andare in pensione un piccolo sacrificio di ulteriore lavoro (ovviamente escludendo i lavori usuranti); ma correggere i coefficienti significa penalizzare ulteriormente quel 35 per cento di pensione che i giovani

so che tanto le questioni che ho posto non avranno risposta. Spero in lei, nel Presidente della Repubblica e nel Presidente della Corte dei conti, per la vostra alta magistratura. Francamente, mi viene in mente Eduardo De Filippo: qui siamo a «Natale in casa Cupiello», dove si spostano le statuine e i pupazzetti, dove si dice: adesso Prodi non va bene, ci mettiamo Veltroni, o Padoa-Schioppa non va bene e ci mettiamo...

è che questo presepio tutto intero non va bene, non le singole statuine, perché non si può poggiare la politica e la politica economica su temi seri come quello delle pensioni, della sanità, del lavoro, della ricerca e dell'innovazione sui falsi in bilancio, sui trucchi contabili, sul dire oggi che c'è e dopodomani che non c'è, a seconda degli equilibrismi (non degli equilibri: magari fossero equilibri) interni ad una maggioranza che non c'è più nel Parlamento, ma soprattutto non c'è più nel Paese. parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà.

la piena delega sull'argomento che stiamo trattando. Questo sarebbe auspicabile, anche perché il contenuto delle due mozioni, quella di maggioranza e quella di opposizione (ma in specie di quella di maggioranza), per alcune parti,

di lunga militanza sindacale e politica, avrà memoria. Correvano gli anni Ottanta e il presidente Andreotti, invitato ad un*panel* di Confindustria nel periodo in cui era presidente

intensità ed entità a causa della riforma Vanoni e del passaggio dall'imposta generale sull'entrata al sistema sul valore aggiunto), ricordò che una volta, quando prima ancora era Ministro delle finanze, aveva ricevuto una folta delegazione di orafi vicentini,

imperitura memoria dell'attenzione del Governo, dichiarato almeno il 20 per cento di quello che fatturavano. Questo succedeva, signor Presidente, nel 1983 o 1984. La situazione è oggi di tutt'altra evidenza; voler considerare, come allora faceva la politica, gli imprenditori, le imprese, gli autonomi, i professionisti come abituali evasori è un atteggiamento proprio

della classe lavoratrice, dei dipendenti subordinati e non autonomi. In un caso bisogna favorire i fattori motivazionali - come dicevamo l'altro giorno - e non quelli igienici e male fa questo Governo a considerare fattore motivazionale l'eliminazione dello "scalone", in quanto quello dovrebbe essere trattato come fattore igienico, mentre maggiore e migliore attenzione dovrebbe essere riservata ai fattori motivazionali come la qualità del lavoro dei dipendenti nell'impresa. assoluta disattenzione in questo momento nell'altro comparto. Quale sia più importante dal punto di vista percentuale non lo sappiamo: emerge da dati statistici e dagli studi di grande rilievo condotti in Europa e nel mondo che i lavoratori autonomi e quelli dell'intrapresa, il popolo delle partite IVA, stanno finendo per

collaborazione leale tra fisco e contribuente e che invece finisce per servire a correggere i comportamenti anomali dei contribuenti, aumentando i ricavi stimati

un significato di sottile ironia: il voler far cadere le mura di Gerico, quasi fossero le mura con cui il contribuente si difende nei confronti dello Stato

se ne riscontrano gli esiti), si ricerca la leale collaborazione del contribuente. Non è possibile alimentare una situazione che è assolutamente inaccettabile, perché il meccanismo operativo che è stato costruito

l'introduzione del sistema sia a valere dal 2007 (richiesta contenuta nella nostra mozione e non già nella mozione di maggioranza). E perché non parlare poi dell'assoluta

tante volte difeso nel corso dell'esame della finanziaria e di altri provvedimenti dal presidente della Commissione finanze, senatore Benvenuto, oggetto delle motivazioni di cui all'approvazione

diceva il senatore Baldassarri, per questi due motivi il Governo dovrebbe essere oggetto di sfiducia, come lo è nel Paese, anche da parte della stessa maggioranza. Come fa, infatti, un Governo a non sapere? Se non lo sa è un Governo inefficiente; se lo sa e non lo dice è un Governo bugiardo

sottolineato a chiare lettere che l'innovazione sostanziale dell'azione del suo Governo, nei confronti dell'azione del Governo precedente, sarebbe stato il rispetto pedissequo e continuo della concertazione con le parti sociali,

se non verrà approvata - cosa che auspichiamo e chiediamo - la nostra mozione, la dichiarazione dei redditi dovrà essere compilata, non tenendo conto delle indicazioni precedenti, ma (per le dichiarazioni dei redditi che già si era cominciato ad elaborare nel mese di aprile) si dovrà tenere conto di una circolare emanata a maggio. Grazie per il fatto che la mozione di maggioranza chiede che non ci sia la maggiorazione dello 0,40 per cento! Ma, benedetto Iddio, c'è bisogno di una mozione per correggere un'attività così vessatoria, così inqualificabile, così

che il gettito non consente di fare a causa di risorse insufficienti. Ma non è vero che le risorse sono insufficienti nel momento in cui si parla di un extragettito che potrebbe rifinanziare di tutto e di più: la spesa sotto controllo sulla sanità; i maggiori trasferimenti agli enti locali; i trasferimenti alle Regioni e - perché no - l'integrazione salariale per il rinnovo del contratto di lavoro per gli statali. Insomma, nel mentre si spende e si spande di tutto e di più, nel mentre il DPEF viene costruito e indicato alle parti sociali ed al Parlamento come un DPEF di rigore e di equità, dal lato della spesa questo non fa che aumentare. Quindi, questa Aula parlamentare dovrebbe fare un decreto, poi recepito dalla finanziaria, per tartassare ancora e di più i cittadini per altri 10 miliardi di euro. Ma per finanziare cosa? Per finanziare la spesa che questo Governo non riesce a trattenere. A questo punto se le stanno inventando tutte: non soltanto con gli studi di settore, ma anche con l'introduzione della tassazione per l'assegno per l'assegno trasferibile rispetto a quello non trasferibile: è su tutti i giornali di oggi, Presidente! Un euro e mezzo per l'emissione degli assegni trasferibili. Ma siamo arrivati al ridicolo, Presidente! Da un lato si dice di poter spendere uno, due, tre, forse quattro miliardi di euro per eliminare lo scalone - imbroglio incluso: se infatti viene mantenuta una quota che va attorno al 97-98 significa che la diminuzione, come ella stessa, Presidente, si è trovato a dire qualche giorno addietro ai giornalisti - non avrà nessun effetto rispetto a quanto richiesto dalla sinistra radicale ed estrema della maggioranza di Governo

sta affossando anche l'Italia. Per questo chiediamo, Presidente, con foga e con convinzione che sia votata la nostra mozione. *(Ulivo)*. Alla luce di quanto è stato detto e di quanto ancora il dibattito potrà dire, mi soffermerò brevemente su alcuni punti nodali che traspaiono dal testo della mozione sottoscritta da alcuni di noi. Vi sono alcuni aspetti da elogiare, su altri devono essere mosse precisazioni. Da elogiare è, senz'altro, una politica fiscale che ha cercato di reintrodurre dei parametri di equità, a fronte di cambiamenti micro e macroeconomici; cambiamenti che tuttavia sollecitano uno sguardo d'insieme a più largo raggio sul mondo del lavoro di cui mai, come in quest'ultimo decennio, si è avvertita una decisa e persistente trasformazione. È chiaro che una realtà frammentata e affatto particolare, com'è quella italiana, con significativi squilibri e disparità nell'ambito del territorio, nonché storicamente fondata su logiche corporativistiche, rende estremamente difficile quando non ardua, la realizzazione di un ampio progetto di riforme: le proteste di alcune categorie in merito al decreto Bersani o le difficoltà di risolvere l'annosa questione dei rifiuti in Campania rappresentano solo alcuni fra i casi emblematici di questi ultimi tempi. Una politica che voglia davvero dirsi riformista è una politica dell'ascolto: capace di instaurare un rapporto virtuoso con la società civile, e dunque con il contribuente. Da qui non si scappa: il quadro generale non può che essere quello di un confronto aperto e costante con le categorie; cosa che fino ad oggi è avvenuta solo parzialmente. In tal senso, gli studi di settore possono costituire un passo in avanti, purché non venga meno la capacità di confronto e di ascolto. Il senso di malessere che si è generato nasce proprio dalle ischemie che si sono create all'interno del sistema di fiducia fra il cittadino e il Governo, non provocando quello scambio e quel confronto che sono gli unici elementi che possono garantire la solvibilità del rapporto. In coscienza, non credo che vi sia oggi una questione settentrionale, ma è doveroso interrogarsi sulle ragioni che sottostanno al malessere che si è creato, in particolare al Nord, perché bollarle con superficialità e pressappochismo sarebbe un grave errore. Tali ragioni sono presto riassunte: gli studi di settore, di per sé, non sono buoni né cattivi. Essi possono essere considerati punitivi solo da chi non ha alcuna intenzione di pagare le tasse. Il problema risiede, semmai, nei parametri ad essi legati. Si limitano a disegnare una griglia, una cartina invisibile che si sovrappone in termini economici alle singole realtà locali. Essi si fondano su una congruità, che deve essere passata al vaglio della coerenza. Ma perché possano rivelarsi strumento utile devono essere uno strumento duttile. La corsa di un autobus, da un capolinea all'altro, non acquista maggior senso nelle ore di punta quando è più affollato: ha lo stesso valore anche nelle corse notturne con pochi passeggeri a bordo. Si muove sulla stessa linea, compie le stesse fermate. Questo tragitto, questa mappa, che altro non sono gli studi di settore, va concordata con le imprese (quelle piccole-medie imprese, non mi si tacci di retorica nel rammentarlo, che hanno fatto negli anni la specificità e la ricchezza dell'azienda Italia), va concordata con il cittadino, con gli utenti. È giusto e opportuno vagliare degli indici di normalità economica, e monitorarne nel tempo le eventuali oscillazioni, senza però perdere di vista le ascisse e le ordinate in cui detta curva variabile si inscrive, che restano congruità e coerenza. La nostra mappa deve avere punti di partenza e di arrivo condivisi, un itinerario certo, fondato su delle regole che non possono essere mutate frettolosamente o *in itinere*, rivedendo dei parametri che si tramutano nei fatti in un aumento puro e semplice del gettito fiscale. c'è un'altra ragione del malessere diffuso su cui è opportuno interrogarsi. Ci vogliono regole chiare, ma anche equità di trattamento. Gli studi di settore costituiscono a loro modo una sorta di sconto per il contribuente virtuoso: se opportunamente regolati sono uno strumento a difesa e tutela degli onesti. In Italia, come ho già detto, non c'è una questione settentrionale: c'è una questione meridionale, purtroppo radicata nella storia del nostro Paese e tuttora lungi dall'essere risolta. E giusto che si vaglino misure adeguate alle singole realtà territoriali, ma è giusto altresì che la tutela degli onesti sia un principio effettivo su tutto il territorio nazionale. Io provengo dall'estremo Nord, da una provincia, ai con la Svizzera, sufficientemente ricca come Varese, e so bene che i micronazionalismi e le culture particolaristiche non portano lontano, rimanendo schiave del malessere che cercano di esprimere. D'altro canto, non posso non domandarmi perché, tutto sommato, sono pochi i parlamentari della maggioranza o dell'opposizione meridionali che abbiano con intensità protestato contro gli studi di settore. Questa è un'anomalia che in qualche modo va sanata, ma va sanata al di fuori dalle logiche, diremo così, ideologiche, metapolitiche o ancor più dalle facili strumentalizzazioni. Una maggiore equità fiscale e il ripristino della legalità non sono patrimonio del centro-sinistra o del centro-destra: sono una moneta buona, un obiettivo da raggiungere. Per tutti, a beneficio di tutti. Non di una parte. Se si vogliono cominciare a gettare le fondamenta di quel Paese nuovo e al passo coi tempi che l'Italia a ragione pretende di essere, è nostro compito fissare un'altezza dell'asticella. Non sarà il Governo a fissarla secondo parametri propri. Dovremo decidere insieme, discutendo con l'opposizione e con le categorie interessate. Fissato il limite, però, non si può più venir meno agli impegni presi, da una parte e dall'altra. Questo è il senso ultimo della mozione in oggetto: stabilire delle regole, instaurare un rapporto di reciproca fiducia con il contribuente entro cui, e non a prescindere dal quale, operare maggiore controllo. Questo significa, secondo giusti princìpi, muovere una lotta costante contro l'evasione e avviare quella politica di riforme dalle fondamenta, di cui mai come oggi, a fronte di squilibri e disparità che si palesano, il nostro Paese ha un urgente bisogno.

ai Ministri, Sottosegretari e personaggi vari che inventano cose come gli studi di settore, ai quali leggo semplicemente uno uno spaccato di vita reale, un articolo apparso qualche mese fa di cui cito i passi essenziali: «Gentile direttore, s*ono un imprenditore metalmeccanico della provincia di Bergamo e la mia azienda impiega otto persone. Lavoro solo per imprese e pertanto tutto quello che faccio è, senza eccezioni, regolarmente fatturato. Grazie agli studi di settore e al decreto Bersani del luglio 2006, quest'anno pagherò, fra tasse e contributi previdenziali, allo Stato l'85 per cento dell'utile conseguito nel 2006. La conseguenza, se non cambiano le leggi, è semplice: sarò costretto a chiudere un'azienda sana, che ha sempre pagato le tasse, dà lavoro a 8 persone e allo Stato non ha mai chiesto niente (per intenderci: mi riferisco a cassa integrazione o prepensionamenti). Ci si può chiedere come faccio a dover pagare l'85 per cento di quello che è il mio guadagno. In realtà, la risposta è molto semplice. Il mio utile prima delle tasse è pari a 98.300 euro. L'utile imposto dal calcolo degli studi di settore, dall'indetraibilità del capannone in cui lavoro (stabilita dal decreto Bersani-Visco del 4 luglio del 2006) è di 139.564 euro. Una bella differenza. Eppure sulla base di questa cifra il totale delle tasse e dei contributi per il 2006 (calcolati appunto sui 139.564 euro di cui parlavo) è di 85.667 euro, ovvero l'85 e passa sull'utile reale. Il bello è che se mi guardo in giro la mia situazione, per quanto possibile, mi appare tutto sommato rosea: alcuni colleghi arrivano a dover pagare anche il 104-114 per cento degli utili che realizzano. Se non ci saranno variazioni a questo sistema di tassazione le conseguenze saranno inimmaginabili. Solo in Lombardia le aziende della subfornitura sono, calcolate per difetto, 90.000, con una media di addetti, sempre per difetto, pari a circa 360.000 persone. La situazione in cui ci troviamo ci impedisce per mancanza di liquidità (dobbiamo pagare più tasse di quello che guadagniamo) di fare investimenti o di assumere personale. In parole povere di far crescere questo Paese.* **Se la situazione non cambia saremo costretti a chiudere.** Per questo motivo ci siamo costituiti in un'associazione». L'articolo poi continua. si tratta di un articolo scritto da un parlamentare leghista o da chissà chi, ma da una persona che potrebbe appartenere a qualunque schieramento politico, che descrive proprio nei dettagli numerici fiscali una situazione che è quella in cui si trova la gran parte delle aziende reali - cioè non quelle statali, pubbliche o assistite - del nostro Paese, in particolare della parte settentrionale Del resto, nella questione degli studi di settore, non a caso inventati ovviamente sempre da personaggi che appartengono al vostro schieramento ideologico, c'è una contraddizione in termini. Lo studio di settore altro un modo per calcolare in maniera automatica e statistica quello che dovrebbe costituire il reddito e di conseguenza la tassazione di un'azienda. Qualche giorno fa Qualche giorno fa il mio capogruppo, senatore Castelli, a proposito della legge sulla sicurezza ha detto che si tratta di una legge scritta da gente che non è mai stata in una fabbrica vera il relatore è un sindacalista, un ex sindacalista (diciamo che dalle nostre parti è quasi la stessa cosa) - e però indicava effettivamente un atteggiamento ideologico, ovvero quello di parlare di questioni che non si conoscono magari si sono studiacchiate sui libri durante il liceo, forse tra un'assemblea e l'altra, tra un corteo e l'altro, finché da grandi si pensa di avere capito tutto della vita. Se una persona normale lavorasse o avesse lavorato e conoscesse da dentro il mondo del lavoro,

Su una serie di parametri che solo la fantasia perversa di qualche cattocomunista può avere inventato: va a vedere il settore merceologico, il consumo della corrente, il numero di addetti, la situazione territoriale, senza immaginare, capire, pensare, o sapere semplicemente, che ogni fabbrica, ogni impresa economica è un ente assolutamente a se stante. Non ci sono due fabbriche uguali, due imprese economiche uguali; a parità di occupazione, di consumo di energia elettrica, di fatturato, quello che ci sta dietro può essere di una differenza abissale. La persona che ha scritto questo articolo è, per è, per dire, una persona che lavora nella subfornitura; in sostanza, sono i terzisti delle aziende più grandi, quelli che danno elasticità ed economia al settore

Non hanno lavoratori in nero perché sono controllati, ma questo è l'ultimo dei motivi perché non lo si fa per principio - è questa la ragione principale - perché non lo si può neanche fare volendo; infatti, quando hai le entrate e le uscite assolutamente registrate, non puoi permetterti neanche un euro in nero perché in automatico diventa utile, come chiunque sia a conoscenza di un minimo di contabilità aziendale capisce immediatamente. Ci può poi essere qualcuno che fa subfornitura, per esempio, per aziende *leader* nel mercato, che fanno prodotti di nicchia, dove magari l'efficacia del servizio è più importante dell'efficienza, cioè del costo, e riescono quindi a spuntare prezzi più grassi. Ci sono altre aziende che lavorano in settori assolutamente maturi, dove la lira al pezzo fa la differenza tra prendere o non prendere il lavoro e, quindi, a parità di fatturato, di consumo di energia elettrica, di persone impiegate, si trovano a guadagnare molto meno. Ci sono aziende che stipulano contratti con prezzi fissati per tutto l'anno, per esempio, con la fornitura della materia prima inclusa nel prezzo; se durante l'anno la materia prima aumenta, qualche volta del 50 per cento, raddoppia o triplica, come succede spesso con le materie plastiche e con i materiali ferrosi, cosa fa l'azienda? benissimo l'anno prima aver guadagnato il 15 per cento del fatturato e l'anno dopo aver perso il 10 per cento. Allora, per voi queste persone che restano attaccate con le unghie e i denti sugli specchi per non chiudere l'azienda, per non mandare a casa gli operai, sono delinquenti? Cioè, voi gli applicate lo studio di settore e devono essere loro a prendersi un avvocato, a far causa allo Stato per dimostrare che lo studio di settore statistico in quel particolare caso non può essere applicato perché non è realistico? È questo l'atteggiamento che voi avete che voi avete nei confronti di queste persone? La vita nelle fabbriche, nei nostri territori, non è questa. È fatta di gente che lavora e paga le

e non va a riparare il rubinetto in casa della pensionata non può evadere le tasse anche volendo. È fisicamente impossibile perché le entrate sono certificate e le uscite devono esserlo altrettanto; se non lo sono diventano automaticamente utile, quindi non si può avere lavoro in nero. Non si può sovrafatturare anche l'acquisto per ridurre gli utili - visto che sicuramente avete la mente perversa - perché, a loro volta, i fornitori sono aziende che hanno lo stesso problema e quindi non possono sovrafatturare. Sono cose normali che dovrebbero sapere tutti, che un personaggio come Visco che arriva dalla Puglia - dove mi pare che l'arte di arrangiarsi rivesta una certa popolarità - sicuramente conosce; conosce; possibile che abbia inventato queste misure per stanare gli evasori, soprattutto quelli delle Regioni settentrionali? Su tutto il resto non vi sfiora neanche il pensiero che magari ci siano altre situazioni da controllare. Ci sono i cinesi, e non solo i 12.000 ufficiali di Milano, ma le centinaia di migliaia che lavorano in nero nei sottoscala o nelle cantine, che questo problema non ce l'hanno, non se lo pongono, non hanno neanche la partita IVA; hanno un ciclo industriale chiuso su se stesso. Abbiamo tutta la miriade di extracomunitari; basta uscire

che appartengono alla normalità; mettetevi nei panni di una persona che mantiene una fabbrica con fatica e dà lavoro a otto famiglie poi alla sera esce stanco dalla fabbrica e mentre va a casa incontra 50 venditori abusivi a cui nessuno dice niente; magari di giorno ha avuto anche la visita della Guardia di finanza che all'andata e al ritorno ha incontrato due volte i 50 venditori abusivi e ogni volta ha girato la testa dall'altra parte. Tuttavia si potrebbero e si dovrebbero dire tante altre cose. L'evasione fiscale per voi cosa è?

E Bassolino, che politicamente li copre e li difende, cos'è secondo voi? Bassolino ha bruciato 2.000 miliardi di tasse, che chiedete alle persone cui applicate gli studi di settore, secondo voi cosa è se non un evasore fiscale? Che differenza c'è tra non pagare una tassa o bruciare in attività inutili quelle che gli altri con grande fatica hanno pagato? Personalmente non ci vedo nessuna differenza, anzi,

nelle aree più calde del Paese da un punto di vista fiscale si porterebbe a casa un grande risultato? Voi vi basate su questo concetto, come anche in altri aspetti: siccome fa fatica andare a scovare chi vive nel nero, oppure pensate di portare a casa grandi quantità di voti in quelle aree oscure del Paese, trovate più semplice andare a beccare chi è già visibile. Pertanto, per ridurre l'evasione fiscale non andate a cercare chi proprio non esiste, cioè i soggetti che non hanno partita IVA, quelli che lavorano in nero, quelli che sono all'interno di filiere industriali completamente nascoste. No, andate a vedere quelli che pagano già e li fate pagare di più. Complimenti, siete veramente dei fenomeni, siete degli statisti! Quindi, andate a beccare l'evasione dove già è più alto il gettito fiscale. Ma io credo che, ad un certo punto, spremere sangue dalle rape, come si dice, sarà abbastanza difficile: alla fine, quando il limone è spremuto lo si può solo buttare via. A meno che quello che voi abbiate in mente è proprio questo. Per cui, se foste onesti intellettualmente, sono tante altre le cose che dovreste andare a guardare. In Italia abbiamo quasi 5 milioni di dipendenti pubblici: mi sembra un po' troppo,

politico-amministrativa. Qualche settimana fa, qualche mese fa, ci sono stati servizi televisivi sui dipendenti della Corte dei conti che entravano in ufficio, ne uscivano dopo un quarto d'ora per andare a fare la spesa, rientravano, timbravano e andavano a casa. Qualcuno di voi è andato a beccare queste persone per vedere perché fanno queste cose, a controllare se lavorano o no e se servono o no? Oppure, stando sempre sui grandi numeri, a nessuno viene mai il dubbio che ci sia qualcosa che non quadra, che ogni volta che cambiano amministratore delegato alle ferrovie dello Stato o all'Alitalia, aziende peraltro che sappiamo producono *cash flow* «di tipo spaziale», ogni volta che la persona fa sei mesi, un anno o un anno e mezzo di lavoro poi lo liquidate con 2, 3, 4 o 5 milioni di euro? Su queste cose nessuno ha niente da dire? Questi soldi, secondo voi, da dove arrivano? Li stampa il Padreterno in Paradiso, poi ogni tanto li manda giù il 27 del mese o c'è qualcuno, su in Padania, che questi soldi - alla fine - li tira fuori? Queste sono tutte cose su cui qualche riflessione profonda, o per lo meno approfondita finché ci riuscite, la dovreste fare. Qualche giorno fa

fa. Ricordo a questo "signore" (non mi viene in mente in che altro modo chiamarlo) che da quando è Primo ministro in questo Paese sono state istituite 60-70 - nessuno le ha contate esattamente - nuove tasse, che alle aziende è stato portato da zero al 10 per cento il contributo fiscale per gli apprendisti, che ai dipendenti è stato aumentato dello 0,3 per cento il prelievo in busta paga, che gli studi di settore - quello di cui stiamo parlando adesso - non contenti di tutto il ragionamento che ha fatto, a marzo sono stati ulteriormente aumentati

ad oggi dal vostro Governo sono solo arrivate tasse in più per le imprese senza neanche un centesimo di euro di riduzione da nessun punto di vista. Questa è la vostra politica dell'immagine, basata sull'annuncio e che vive di ideologia.

Voi avete in mente un Paese composto solo da gente che ha in tasca la tessera del partito, del sindacato, della Coop o di qualcos'altro e vi vota, mentre tutti gli altri sono evasori: peccato che questi evasori paghino le tasse che pagano anche il vostro stipendio.

innanzitutto a questa maggioranza il fatto ed il merito di aver per prima dato ascolto alle legittime richieste delle rappresentanze delle piccole e medie imprese, e per prima di aver segnalato al Presidente del Consiglio dei ministri, con una lettera del 13 giugno scorso, d'iniziativa della sottoscritta e condivisa anche da altri colleghi, la necessità di correggere l'azione dell'amministrazione finanziaria sulla gestione degli studi di settore ed in particolare dei nuovi indicatori di normalità economica, mentre l'opposizione era ancora

dell'azione del Governo e della maggioranza. La nostra azione politica e la nostra mozione sono coerenti anche con quanto abbiamo dichiarato nella discussione della manovra finanziaria per il 2007. L'attuale maggioranza, avendo la consapevolezza di dover operare un rapido ed incisivo risanamento della situazione dei conti pubblici ereditati, si è assunta la responsabilità di approvare una manovra che per poter dare risultati nel breve periodo di un anno agisse prevalentemente sul lato delle entrate, rinunciando a proporre emendamenti a proporre emendamenti al decreto fiscale collegato alla finanziaria, ma presentando degli ordini del giorno, considerati impegnativi d'intesa con il Governo, con il Governo, che impegnavano in sostanza l'Esecutivo a realizzare finalmente i presupposti di un nuovo patto tra fisco e contribuente, da un lato, con l'impegno a destinare le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale alla riduzione della pressione fiscale raggiunta nel 2007, dall'altro, richiamando la necessità dì dare piena attuazione e rispetto ai contenuti dello Statuto del contribuente. Ebbene, gli obiettivi di risanamento che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti, ma non possiamo dire altrettanto degli impegni che il Governo si era assunto con la sua maggioranza in ossequio a quegli ordini del giorno. Come ha rilevato il Governatore della Banca d'Italia nella sua recente relazione annuale: «il recente miglioramento dai conti pubblici è dovuto - soprattutto - al forte aumento delle entrate e le stime del Governo indicano per quest'anno un ulteriore incremento della pressione fiscale. Il livello è più alto della media europea; è prossimo ai massimi degli ultimi decenni. Le aliquote legali delle imposte che gravano tanto sul lavoro quanto sul capitale sono elevate» - per cui, conclude il Governatore: «livello eccessivo del prelievo, variabilità e complessità delle regole fiscali scoraggiano l'investimento in capitale fisico e umano e rendono più onerosa l'osservanza delle norme». Dunque, se era accettabile - per i motivi che ho detto - nel breve periodo un risanamento basato in gran parte sull'aumento dell'entrate, ora, visti i risultati della manovra finanziaria e l'attuale livello della pressione fiscale, se vogliamo che il Paese torni a crescere in modo continuativo, dobbiamo sostenere di più chi produce ricchezza e non asfissiare la realtà produttiva del Paese con ingiustificati aggravi di adempimenti e ulteriore allargamento di base imponibile. È giunto il momento di dare un forte segnale, sia sul versante del miglioramento della qualità e produttività della spesa pubblica, sia di alleggerimento del carico fiscale sui milioni di imprese e lavoratori che ogni giorno rischiano e si confrontano, senza ammortizzatori, con il mercato e la concorrenza. Bisogna cioè rendere contestuale il recupero di base imponibile (ottenuto attraverso la lotta all'evasione e all'elusione fiscale) con la riduzione del prelievo fiscale su coloro che lavorano e producono ricchezza per il Paese, contrastando piuttosto le rendite di posizione. Sarebbe controproducente per la missione di crescita che vogliamo per tutto il Paese contrapporre l'interesse dei lavoratori dipendenti con quello dei lavoratori autonomi e degli imprenditori. Entrambi chiedono allo Stato di spendere meglio le risorse della fiscalità generale, entrambi chiedono all'amministrazione finanziaria di essere più incisiva non solo nel denunciare, ma anche nello stanare gli evasori, soprattutto i grandi evasori, perché tutti i contribuenti leali ritengono di pagare tasse troppo alte per il livello dei servizi pubblici che vengono loro erogati. E sono convinta che solo uno Stato che si preoccupa di salvaguardare, accanto al lavoro dipendente, anche l'equilibrio economico delle imprese, solo quello Stato può raggiungere obiettivi di crescita e sviluppo ed insieme di equità sociale. Per questo la nostra mozione è volutamente più ampia, e non si limita alla sola questione dei nuovi indicatori di normalità economica, che costituiscono un aspetto importante, ma non esaustivo dei correttivi alla politica fiscale del Governo di cui oggi il Paese ha bisogno. L'azione che la maggioranza ha promosso per prima in ordine agli studi di settore ha avuto comunque un riflesso politico importante. È significativo che a Treviso, durante la manifestazione di protesta di artigiani e commercianti di sabato scorso, fosse stato affisso uno *slogan* che recitava, più o meno: «Pagare le tasse è un dovere. Chi evade è il primo nemico delle imprese. Vogliamo un fisco con regole certe ed eque». Credo che questo *slogan* sia un segnale importante della possibilità di dar vita ad un nuovo, costruttivo rapporto anche tra fisco e piccole imprese, fondato sulla legalità e ragionevolezza, segnale che il Governo deve dimostrare con i fatti di saper cogliere, dopo anni ed anni di sanatorie e condoni che hanno favorito l'evasione fiscale, quando non è stata addirittura incoraggiata dalle stesse parole dell'allora *Premier* ed ora capo dell'opposizione. Ci aspettiamo dunque un immediato, concreto, segnale dal Governo di riapertura del dialogo con le rappresentanze di categoria, di rispetto scrupoloso delle norme e dei princìpi dello Statuto del contribuente, a cominciare dall'applicazione concertata e non retroattiva degli studi di settore e dei nuovi indicatori di normalità economica, sulla base dei quali non è ammissibile alcun automatismo accertativo a favore dell'amministrazione finanziaria e tantomeno alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. A questo proposito vorrei ricordare ai colleghi dell'opposizione che la giusta rivendicazione delle categorie di cui parliamo oggi assomiglia a quella che era stata promossa nell'aprile dello scorso anno delle stesse categorie, dopo che con un decreto-legge del 10 gennaio 2006 il Governo Berlusconi aveva spostato al 2 maggio il termine del 31 marzo Presidente della Repubblica n. 195 del 1999, debbono essere pubblicati i decreti contenenti i nuovi studi di settore per poterli applicare al periodo d'imposta dell'anno precedente. Anche allora venne giustamente affermata la violazione dell'articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente, il che dimostra che il problema di un fisco più giusto e più equo è un problema che in questo Paese va ben al di là delle singole maggioranze e dei singoli Governi. Perciò nell'affrontare tematiche di questo spessore e nel tentare di cogliere le ragioni di un malessere sociale, vogliamo oggi, con la nostra mozione, riaffermare i princìpi di giustizia fiscale che devono informare il nostro sistema. Tra questi, quello di capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione), il quale impone al legislatore di adattare i modelli di prelievo al singolo contribuente e non alla massa, e le norme dello Statuto del contribuente, definite «quasi costituzionali» dalla giurisprudenza dellaCassazione. Credo, e mi avvio alla conclusione, che in attuazione di questi princìpi di buona fede e affidamento e di divieto di retroattività, sia la stessa revisione postuma degli studi di settore consentita dal predetto decreto del Presidente della Repubblica del 1999 che andrebbe eliminata. Gli studi di settore dovrebbero essere approvati entro marzo dell'anno di competenza e non dell'anno successivo, in modo da persuadere i contribuenti sleali a modificare nel corso dell'anno il loro comportamento scorretto. Gli studi di settore tornerebbero così alla loro funzione principale di strumento preventivo e dissuasivo dell'evasione, e non repressivo. Su questo mi riservo, con altri colleghi, di valutare una conforme modifica legislativa. Il rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria è uno degli indici con cui si misura la civiltà del diritto di uno Stato. Il rispetto delle regole, come vale per il contribuente, deve valere anche per il fisco, che non può pretendere di cambiarle in corso d'opera. Ci aspettiamo perciò che il Governo conformi da subito la sua azione e quella dell'amministrazione finanziaria al preciso mandato che oggi la maggioranza che lo sostiene esprime con la mozione in oggetto.

signor Sottosegretario, accolgo con piacere dalla senatrice Rubinato la notizia che lei non ha più la fiducia della sua maggioranza, così

sono talmente vicini a quelli del centro-destra da farci pensare che la mozione presentata dal nostro presidente Schifani stata così ampiamente condivisa da aver contaminato anche la maggioranza di questo ramo del Parlamento, che evidentemente

spesso particolarmente ostile alla popolazione italiana di uno dei ministri più in vista del suo Governo, cioè del ministro Visco). vorrei anche ricordare alla senatrice Rubinato che quel presidente Berlusconi del quale ella parla a proposito del presunto invito ad evasione fiscale è lo stesso Presidente del Consiglio che invece, unico nella storia del nostro Paese, è riuscito a fare incrementare nell'arco di pochi anni, con una politica fiscale di segno esattamente opposto a quella incarnata dal vice ministro Visco, il gettito erariale e le entrate fiscali.

pubbliche, che - occorre ricordare sempre più spesso - sono proprio quelle che arrivano dalle tasche degli italiani, di tutti gli italiani, di coloro che pagano le tasse ovviamente, vi servite di quelle risorse per finanziare e sostenere iniziative e scelte politiche quanto mai opinabili, alcune delle quali sono state ampiamente ricordate in quest'Aula. Esse parrebbero più premiare aree più premiare aree culturali e lavorative del nostro Paese di tipo assistenzialistico piuttosto che sostenere gli sforzi continui che tanti lavoratori autonomi, tanti professionisti, tanti piccoli e piccolissimi imprenditori, artigiani e commercianti fanno ogni giorno per garantire al nostro Paese un gettito erariale che è di tutto rispetto. La riforma degli studi di settore che è oggetto della nostra mozione - vale la pena ricordarlo - fu attuata all'insegna di meccanismi automatici che allora avevano l'effetto di riportare l'Italia in quella media europea di gettito fiscale. La vostra riforma, quella che presentate per per iniziativa del vice ministro Visco, invece, non solo è attuata all'insegna di meccanismi automatici decisi unilateralmente dal Governo senza nessuna consultazione con le parti, ma ha sortito già degli effetti paradossali, ovvero invece di fare emergere nuovi contribuenti, ha brutalmente raddoppiato il numero delle aziende che oggi non sono più in grado di essere considerate, secondo il frasario ed il linguaggio degli studi di settore, congrue.

e però conferma un dato, cioè che chi era evasore lo è rimasto e nulla è stato immaginato per aumentare quei controlli che possano aiutarci a fare emergere il lavoro sommerso, il lavoro nero e tanta economia nera del nostro Paese che che sottrae (è stimato dai dati dell'OCSE) circa il 25 per cento del nostro PIL ufficiale. Nel protocollo stilato tra il vostro Governo e le associazioni di categoria a dicembre c'era un passaggio molto importante: quell'accordo di Natale aveva come finalità la diminuzione del numero delle imprese non congrue e non certo il suo raddoppio, come invece è già avvenuto. Vorrei poter allontanare da tutti noi il rischio di facili demagogie da una parte, ma anche dall'altra, ed è opportuno soffermarsi brevemente sulle ragioni che hanno indotto il legislatore ad inserire gli studi di settore nel nostro sistema fiscale. Le motivazioni furono le più eterogenee, riconducibili innanzitutto al sospetto di evasione dei piccoli imprenditori, alimentato, a sua volta, da scarsa credibilità dei dati dichiarati, ora all'eccessivo garantismo delle scritture contabili, ora alla oggettiva difficoltà dell'amministrazione finanziaria di argomentare e motivare avvisi di accertamento incentrati sulla valorizzazione di elementi extracontabili. Sicuramente l'intento del legislatore era quello di reagire a fattispecie evasive delle quali si ha una forte percezione e per le quali tuttavia è difficile passare all'azione, setacciando una platea di contribuenti vastissima e scovando, all'interno di questa, i singoli responsabili. Tuttavia, con l'ultima riforma Visco-Bersani si è andati oltre quanto era lecito aspettarsi, trasformando gli studi di settore da mero strumento presuntivo di accertamento ad uno strumento

essenzialmente svolgere una funzione di orientamento nella selezione dei contribuenti da controllare, utilizzando a tal fine il criterio della grave incongruenza tra il reddito dichiarato dal contribuente e quello presunto sulla base della stima del reddito medio di settore di attività. Pertanto, lo studio di settore deve rappresentare, vista la sua natura presuntiva, solo un mero strumento di accertamento e non un criterio di automatica quantificazione della materia imponibile. Se così non fosse, infatti (come da più parti ricordato, persino dalla senatrice Rubinato), verrebbe violato il principio di capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione, in quanto l'individuazione dell'indice di disponibilità di mezzi economici per far fronte al riparto delle spese pubbliche avverrebbe sulla base non non già del reddito effettivo, ma di un reddito riferibile ad una pluralità di soggetti e, dunque, determinato sulla base di elementi riconducibili alla "normalità", alla "massa", non alla singola capacità e responsabilità. II principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione impone una personalizzazione della contribuzione, dovendo avere riguardo all'effettività dell'arricchimento; diversamente, gli studi di settore si basano su schemi impositivi di natura matematico-statistica, prescindendo dal riferimento alle scritture contabili che, invece, rappresentano la regola nella determinazione del reddito effettivamente prodotto. Alla luce di tali considerazioni deve essere mutata la posizione dell'amministrazione finanziaria, espressa nella circolare del 22 maggio 2007, n. 31/E, secondo cui la modifica introdotta dal decreto Visco-Bersani agli studi di settore non ha altra finalità se non quella di ribadire la valenza probatoria dei ricavi e dei compensi stimati sulla base dello studio di settore. Di talché l'accertamento basato sugli studi di settore può essere effettuato ogni qualvolta il contribuente dichiari ricavi o compensi non congrui rispetto alla stima, senza che l'amministrazione finanziaria debba fornire ulteriori dimostrazioni a sostegno della pretesa tributaria. Anzi, come ben sapete, è il cittadino contribuente che deve difendersi dalla presunzione dello Stato, il quale gli affibbia un reddito che magari non riesce Ciò è del tutto inaccettabile. In questo modo il dato matematico-statistico su cui si basa lo studio di settore si sostituisce al dato risultante dalle scritture contabili: la massa si sostituisce al singolo, inserendo un elemento normale nella base imponibile che, in virtù delle scelte effettuate sul versante sostanziale, dovrebbe invece essere connotata da analiticità e da effettività. Inoltre, la constatazione che gli studi di settore colpiscano esclusivamente i piccoli imprenditori e tutti quei soggetti economici che ho citato prima conduce al paradosso secondo cui solo per questi e per coloro che si trovano in questa situazione i dati risultanti dalla contabilità non corrispondono necessariamente alla sostanza reddituale e che tale scarto debba ricomporsi per via statistica. Mi pare una discriminazione decisamente insopportabile. In conclusione, gli studi di settore, pur rappresentando uno strumento di immediato incremento del gettito erariale, nonché di contrasto a fenomeni evasivi, non può esonerare l'amministrazione finanziaria dalla dimostrazione che i risultati reddituali derivanti dall'applicazione dello specifico studio di settore siano concretamente riferibili allo specifico contribuente sottoposto a controllo, nel rispetto così di princìpi di giustizia sociale ed economica. Noi auspichiamo quindi una immediata correzione da parte del Governo, non solo perché quella retroattività è sembrata odiosa a chiunque, ma perché questo Governo deve comprendere che, vista la mozione illustrata dalla senatrice Rubinato, non ha più il sostegno nel Paese e nemmeno in quest'Aula, anche se in questo momento è così vuota. ha l'obbligo di comprendere soprattutto che alzare l'asticella delle tasse sulla base delle necessità di cassa non significa rispettare gli studi di settore. Gli studi di settore sono uno strumento che, come abbiamo dimostrato, hanno una loro utilità. Certo, non rispondono a quella visione romantica che ne ha dato il senatore Rossi prima, ma sono comunque uno strumento di controllo, che voi rischiate di trasformare in uno strumento di controllo poliziesco. Altro che lotta all'evasione fiscale!

Il Protocollo che questo Governo ha sottoscritto con le categorie, per poi ingannarle qualche mese dopo, parlava chiaro: gli indicatori dovevano essere concordati con le associazioni di categoria. Al suo vice ministro Visco, signor Sottosegretario, che conferma ancora una volta la sua triste fama di «Dracula, presidente dell'AVIS», consigliamo di rimangiarsi tutto e di ripartire da lì. *(Applausi

finestra") *(Aut)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, la mozione presentata dalla maggioranza e predisposta con un nostro notevole contributo contiene l'impegno a dare seguito a quanto previsto nel DPEF 2007-2011, approvato nel luglio 2006. Il riferimento è riportato letteralmente nella mozione, e chiedo di poterlo allegare Ciò che chiediamo con la mozione è proprio la realizzazione di quanto questo programma prevede per evitare che rimanga un libro dei sogni. Diamo un segnale ai cittadini di coerenza e credibilità, un segnale tangibile e concreto: fatti e non solo promesse. In particolare, con la mozione chiediamo di allineare la politica fiscale a quella degli altri Paesi europei, e cioè evitare norme fiscali con effetti retroattivi, dando così certezza di diritto ai cittadini, nel rispetto dello Statuto del contribuente; diminuire ragionevolmente gli obblighi burocratici e, in particolare, esonerare dall'obbligo di presentazione dell'elenco clienti-fornitori, per il 2006, i piccoli imprenditori e gli esercenti arti e professioni; venire incontro alle categorie per quanto riguarda le scadenze dell'invio telematico delle dichiarazioni; creare uno spirito di collaborazione e di confronto sereno tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti; effettuare controlli mirati per combattere efficientemente l'evasione fiscale e, di seguito, arrivare ad una riduzione della pressione fiscale per tutti i cittadini.

tutte le garanzie ai contribuenti circa il fatto che lo studio di settore non costituisca una *minimum tax*; deve essere invece un punto di partenza per un confronto fra l'amministrazione e il contribuente. Questo concetto vorrei fosse ancora ribadito per tutti coloro che hanno dei dubbi. Ci deve essere un confronto sereno e corretto tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente su documenti contabili e situazioni reali; dobbiamo garantire che le tasse si pagano sui redditi effettivi e non su redditi fittizi imposti. Ma stiamo attenti, perché con gli indici di normalità economica si vanno a colpire le attività minime e marginali, prevalentemente le attività dei giovani, degli anziani e delle donne. Pertanto, come affermiamo nella mozione n. 114, gli indicatori di normalità economica individuati con il decreto ministeriale 20 marzo 2007 devono avere natura sperimentale, devono essere utilizzati secondo il Protocollo firmato dalle categorie nel dicembre scorso per formare le liste selettive di controllo e non devono assolutamente dare avvio ad accertamenti automatici. Si intende poi, naturalmente, che nei controlli l'onere della prova rimane a carico dell'amministrazione. Signor Presidente, sono soddisfatta per il fatto che grazie ai nostri interventi svolti nelle Commissioni e, infine, qui in Aula siamo riusciti a determinare un'inversione di rotta della politica fiscale del Governo allineandola, con l'approvazione di questa mozione, agli obiettivi da noi previsti nel DPEF 2007‑2011 più volte citato. La nostra mozione infatti va nella direzione giusta: dà le risposte alle fondate preoccupazioni dei contribuenti e imposta la politica fiscale sui princìpi di equità, di sviluppo, di semplificazione degli adempimenti per arrivare ad una progressiva ma effettiva riduzione della pressione fiscale per tutti i cittadini. Ci aspettiamo che con l'approvazione della mozione vi sia l'impegno politico del Governo e della maggioranza di prevedere norme *ad hoc* già nel prossimo disegno di legge in materia fiscale che sarà esaminato in quest'Aula a partire dai prossimi giorni. Dobbiamo dare ai cittadini certezza e prospettive.

prendo brevemente la parola per precisare un importante aspetto affrontato nella mozione di maggioranza nelle more di dare voce

mie considerazioni erano in un punto proprio del considerato; mi riferisco alla parte in cui si fa riferimento al necessario aggiornamento e revisione degli studi di settore. Ben più opportuno sarebbe stato l'inserimento di tale rilievo nel dispositivo della mozione stessa proprio al fine di dare certezza a quello che pare sia l'intento del Governo ossia affrontare nell'immediatezza l'indispensabile revisione degli studi di settore, previa concertazione con tutte le categorie economiche interessate. Ma nell'impossibilità dettata del Regolamento di poter procedere ad una modifica della mozione in tal senso, vorrei comunque avere indicazione dal sottosegretario Lettieri, che in questo momento è distratto. Mi scusi,

dei tempi precisi e ravvicinati per dare avvio a quel tavolo di concertazione fondamentale affinché il processo di definizione della mozione sia più chiaro a tutti.

l'autorizza in tal senso. GIARETTA *(Ulivo)*. Mi limito solo ad una brevissima considerazione. La nostra richiesta di correzione sulle politiche fiscali del Governo nei confronti delle piccole imprese e del lavoro autonomo - perché di questo si tratta di questo si tratta - naturalmente non si applica sul punto della lotta all'evasione né sulle buone e necessarie manutenzioni degli strumenti che lo sorreggono. Il punto è un altro: una efficace politica di lotta all'evasione non può realizzarsi senza un livello adeguato di consenso con chi è intermediario tra il fisco e il contribuente, il sistema delle attività professionali e la realtà dell'associazionismo economico. Credo di conoscere abbastanza bene il mondo delle associazioni del lavoro autonomo. Sono una parte importante dell'organizzazione della democrazia sostanziale del nostro Paese. Non luoghi di organizzazione dell'evasione fiscale, ma piuttosto di formazione alla imprenditorialità, di aiuto alla crescita organizzativa delle imprese, di cooperazione, di organizzazione di forme avanzate di democrazia economica; se serve, anche di accompagnamento all'uscita dall'area della marginalità dell'evasione del lavoro nero. È essenziale, perciò, un rapporto positivo con queste organizzazioni. Sappiamo che c'è uno strumento per tornare ad un rapporto positivo. È il protocollo del 14 dicembre. A quel protocollo dobbiamo tornare perché prevede una serie complessa e coerente di adempimenti condivisi e di reciproci impegni. È stato un errore discostarsi da quel percorso. È un errore che è possibile correggere. La mozione della maggioranza invita con chiarezza a farlo. Rivedere le proprie decisioni di fronte ad argomentazioni fondate non è mai un segno di debolezza della politica. È semmai un segno di saggezza. Siamo certi che il Governo darà adempimento con convinzione agli orientamenti del Parlamento.

interesse e puntualità, anche quelli molto critici nei confronti del Governo e che hanno magari un'altra visione

cittadini italiani, fortemente impegnati nella crescita del nostro Paese, quali sono gli artigiani, i commercianti, i piccoli imprenditori, i liberi professionisti e così via.

che i bilanci, i conti pubblici presentati da questo Governo e faticosamente messi in ordine sono trasparenti. potrà discuterne certamente - ed è diritto del Parlamento e dovere del Governo presentare conti veritieri - e l'occasione prossima è quella dell'assestamento di bilancio e del DPEF. Quindi, nessun problema per quanto riguarda questo

e favorì molto gli investimenti nel nostro Paese. È vero che andava più nella direzione del sostegno alle imprese maggiori, ma portò a risultati notevoli. Quegli sono dati facilmente rintracciabili.

Credo che il Paese sia unanimemente impegnato a guardare ai problemi della crescita economica e a mettere da parte le tentazioni di tipo assistenzialistico. Non dimentichiamo però che anche la solidarietà per cui dobbiamo attivare e adottare politiche di ausilio per coloro che sono rimasti indietro. Questo fa parte della nostra cultura, non solo di noi che stiamo al Governo, ma credo dell'intero popolo italiano.

ma strumenti statistici relativi all'attività dei lavoratori autonomi e dei professionisti. Voglio ricordare che furono costituiti sulla base delle informazioni fornite dagli stessi contribuenti in relazione alla propria attività, secondo le le diverse tipologie dimensionali, settoriali e territoriali. Gli studi, mi preme sottolinearlo, furono sottolinearlo, furono concordati, nacquero in accordo con le categorie per superare le ingiustizie - ve lo ricorderete - e le rigidità della *minimum tax*

anche una sorta di sconto. Vorrei ricordare questo aspetto. Se i lavoratori autonomi, le piccole imprese e i professionisti che guadagnano, per loro fortuna e per loro capacità,

e, allo stesso tempo, un supporto all'Agenzia delle entrate nella predisposizione delle attività prioritarie di accertamento. Il senatore Galli ha ricordato che devono essere semplicemente uno strumento di riferimento per l'amministrazione nel decidere l'accertamento; concordo e condivido pienamente, perché l'accertamento non è automatico. Questa è la genesi degli studi di settore. I Governi che dal 1993 si sono succeduti li hanno considerati tutti utili; non soltanto il Governo che allora decise di istituire tali studi, ma anche quelli che si sono succeduti e alternati nel tempo. Voglio ricordare ancora che le stesse categorie degli artigiani e dei commercianti non ne hanno mai contestato la validità. Quindi, sono uno strumento accettato. Non consideriamo gli studi di settore una *minimum tax*, né la catastizzazione dei ricavi dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese. In merito, voglio precisarlo in maniera molto limpida, la posizione del Governo è la seguente. Si ribadisce che gli studi di settore non sono il Vangelo, come ho detto precedentemente, e quindi deve essere chiaro, non solo agli onorevoli senatori ma anche alle categorie professionali e agli uffici dell'amministrazione finanziaria, che il contribuente autonomo, come tutti gli altri, se da un lato ha il dovere di dichiarare il reddito reale, non ha però l'obbligo di adeguarsi al livello di congruità indicato nello studio di settore a lui applicato. Se l'artigiano, il commerciante, il professionista, la piccola impresa ritengono che il livello di congruità dello studio non rispecchi la loro specifica realtà di impresa e di lavoro, essi non sono tenuti ad adeguarsi. Questo è l'orientamento, la volontà, la decisione ufficiale del Governo.

scaturisce non da un'azione generosa del Governo, ma dal fatto che se da un lato c'è il dovere di lottare contro l'evasione, dall'altro c'è anche l'obbligo di rispetto verso il contribuente, il contribuente, prioritario rispetto a qualsiasi altro obbligo. Un obbligo che ci deriva da una profonda convinzione, oltre che da un obbligo di legge qual è lo Statuto del contribuente, su cui, detto onestamente (non vi sembri una provocazione), qualche violazione nel corso degli anni da parte di tutti i Governi vi è stata con la famosa retroattività. Chi vi parla nel quinquennio scorso sedeva nei banchi dell'opposizione e mosse, come avete fatto voi, amici senatori dell'opposizione, critiche all'allora Governo per avere violato lo stesso principio. È capitato purtroppo anche a noi, data l'anomala situazione economica nella quale ci siamo venuti a trovare, di valutare un elemento che non sempre è stato rispettoso dello Statuto del contribuente, che, ripeto, va comunque rispettato. Da oggi in poi certamente si farà del tutto perché non vi sia più applicazione di questa retroattività. La lotta all'evasione e all'elusione fiscale, su cui il Governo è fortemente impegnato, mira però anzitutto a scovare gli evasori totali, a colpire le società cartiere, quelle che nascono soltanto per emettere fatture false o quelle che illegalmente hanno o gestiscono fonti nei cosiddetti paradisi fiscali. Voglio ricordare che questa volontà di lotta all'evasione è partita dal primo momento in cui si è insediato il Governo Prodi, dicendo che non avremmo fatto più condoni. Senza amor di polemica, voglio ricordare che il condono relativo agli anni 1998- 2002 fatto dal precedente Governo purtroppo è stato un pessimo segnale. avrà pure fatto aumentare le entrate in quel periodo ma, unito soprattutto allo scudo fiscale, con un regalo del 2,5 per cento a coloro che avevano esportato illegalmente capitali all'estero, è stato un messaggio devastante anche per i contribuenti onesti. L'ho voluto ricordare non come un fatto di polemica ma per dire che nelle attività legislative e governative non sempre si riesce ad essere davvero coerenti con le dichiarazioni programmatiche che il Governo presenta al Parlamento. Per quanto riguarda il condono previdenziale per gli agricoltori, più che un condono è una rateizzazione dinanzi ad una difficoltà dell'agricoltura non lo dimentichiamo, è ancora il settore primario - che ha una esposizione debitoria. Vedo qualche senatore meridionale che conosce molto bene la situazione di dramma che vivono gli agricoltori, i produttori ortofrutticoli della Sicilia, della

Comprendiamo il ruolo dei professionisti, dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese, intendiamo ripristinare

augurandoci e sforzandoci che vengano superate le rigidità e le incomprensioni che vi sono state, probabilmente, se volete, anche per sottovalutazione dello stesso Governo. In tal caso, mi assumo per intero la mia responsabilità. Sono convinto che una politica fiscale più equa e semplice possa essere insieme agli operatori professionisti e alle stesse categorie nell'interesse dell'intero Paese e dell'economia italiana. Esprimo parere

anche se - voglio dirlo con franchezza - al di là della critica netta che c'è alla politica del Governo, qualche passaggio potrebbe al limite essere condivisibile, ma ritengo sia già contenuto nel testo della mozione presentata dalla maggioranza.

pressione fiscale per le famiglie e le imprese, nonché di riduzione delle imposte sulla prima casa

Avendo stabilito nella Conferenza dei Capigruppo che comunque si procede al voto degli strumenti che sono stati presentati, mi vedo costretto ad armonizzare i tempi delle dichiarazioni di voto

Signor Presidente, i primi saranno gli ultimi, non gli ultimi saranno i primi. PRESIDENTE. Così scrivevano anche in testi ben più importanti. Signor Presidente, colleghi, quest'oggi il Parlamento responsabilmente fa sentire la sua voce sui temi caldi della politica fiscale del Governo e intende farlo segnando un impegno chiaro per l'Esecutivo, che dovrà trovare immediata concretizzazione. Fino a questo momento il Governo ha mostrato un atteggiamento di forte chiusura, attestandosi su posizioni irremovibili e suscitando un malcontento diffuso; occorre adesso dare invece un segnale altrettanto forte al Paese, recuperando la frattura che c'è stata con l'opinione pubblica su un tema delicato per i cittadini come quello dell'imposizione fiscale. Come potrebbe altrimenti mantenere fermo il proposito, espresso nel programma nel programma presentato alle Camere, di voler costituire un rapporto amichevole tra cittadini, imprese, famiglie e Fisco? La soluzione invocata per il bene del Paese, per combattere realmente la lotta all'evasione fiscale e al sommerso, non è certamente quella di un rigore fiscale fine a sé stesso. C'è necessità di dare anzitutto ascolto e voce agli addetti ai lavori, alle associazioni di categoria, alle parti sociali e la maggioranza di questo ramo del Parlamento, attraverso la mozione che stiamo discutendo, compie un passo decisivo in questa direzione. C'è necessità di ricerca di soluzioni immediate, che siano concertate e condivise; c'è necessità di superare definitivamente le violazioni palesi dello Statuto del contribuente che si stanno perpetrando attraverso l'adozione di misure retroattive, come quella per cui gli indicatori di normalità economica, introdotti con la finanziaria per il 2007, che debbono essere applicati per le dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 2006. È per questo che vogliamo impegnare il Governo a consentire l'applicazione in senso sperimentale di tali indicatori: come è possibile che non ci si renda conto delle scadenze operative incombenti e che, date le evidenti difficoltà nell'applicazione della suddetta normativa, si pongano in essere soluzioni tampone, come la grottesca proroga di termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, quando invece non si ha la benché minima certezza circa i parametri da utilizzare per redigere le dichiarazioni stesse? Sarebbe meglio aprire gli occhi e osservare le certezze tangibilissime che balzano in maniera lampante: l'esigenza l'esigenza di poter procedere nel più breve tempo possibile alla rivisitazione negli studi di settore, coinvolgendo da subito tutte le categorie interessate; l'esigenza di posticipare la scadenza per l'invio telematico del modello unico al 30 settembre; l'opportunità di revisione dell'obbligo di presentazione dell'elenco dei clienti e dei fornitori e l'esonero delle realtà produttive più piccole. sono i contenuti fondamentali della mozione che i Popolari-Udeur intendono sostenere con fermezza, convinti più che mai che si debba cambiare uno *status quo* che sta mettendo in seria difficoltà migliaia di aziende: ricostituire un rapporto costruttivo con le associazioni di categoria e fornire un sistema di norme certe, nell'obiettivo fondamentale della lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Come dicevo, noi dell'Udeur

ci stanno ascoltando e debbono sapere che il Governo non c'è. Loro non possono vedere, però io devo testimoniare che, e non soltanto per questo argomento (anche se peraltro devo dire che ‑ insisto ‑ la sua presenza non è stata di quantità, ma di qualità), si è trattato di una presenza insufficiente a giustificare un'azione inesistente, rispetto ad una richiesta del Senato, peraltro concordata unanimemente in Conferenza dei Capigruppo.

però, fra di noi c'è chi questa difesa la farà ad oltranza. Chiedo scusa per la divagazione, necessaria a dimostrare in quale clima siamo costretti a lavorare. L'opposizione si rende qui oggi portatrice delle molteplici e forti proteste che si sono sollevate dalle categorie produttive del Paese, critiche che non sono mai mancate, ad onor del vero, dall'insediamento di questo Governo e dal compimento dei suoi primi atti di politica fiscale e di lotta all'evasione, come dicono. Ad accendere questa miccia, ultima solo a livello cronologico, è stato l'ennesimo tentativo di introdurre surrettiziamente un inasprimento della pressione fiscale a scapito dei contribuenti e degli onesti lavoratori che le tasse le pagano. La preoccupazione è alta in tutto il Paese e la contrarietà, rispetto al sentiero intrapreso dalla finanziaria di quest'anno, si manifesta oggi in un accorato grido contro gli studi di settore, divenuti arma brandita in modo unilaterale da questo Governo per minacciare, punire, opprimere il povero contribuente soffocato dalle tasse e dagli adempimenti burocratici sempre più cavillosi e impraticabili, disattendendo lo stesso accordo firmato, con i ministri Bersani e Visco, dalle Associazioni nazionali dell'artigianato e del commercio nel dicembre 2006. Le organizzazioni di settore denunciano la non funzionalità di questo strumento, la difficoltà di segnalare le anomalie, che conduce solamente ad introdurre un ulteriore livello di tassazione che incide sui liberi professionisti, sulle piccole imprese, ma soprattutto sui giovani, i quali dovrebbero essere esonerati dall'applicazione degli studi di settore per facilitarne l'introduzione nel mercato. Siamo stati capaci di sognare i sogni: anche questo è da mettere nel *carnet* dei vostri primati. Gli indicatori, attualmente, così previsti, a opinione comune e della stessa Confindustria, si traducono inevitabilmente in una pressione fiscale slegata dalle attività reali delle imprese. La Casa delle Libertà con la nostra mozione chiede inoltre al nostro dissennato Esecutivo di eliminare ogni effetto retroattivo sui redditi del 2006, per poter in qualche modo ovviare ai danni causati alla nostra economia. Ciò che ormai non desta stupore, ma solo amara ilarità, sono le azioni messe in campo negli ultimi giorni dalla stessa maggioranza, che ancora una volta corre ai ripari per ovviare ad un pasticcio del suo Governo, da essa stessa avallato al momento dell'approvazione della finanziaria. Ma al pasticcio si aggiunge, come al solito, un altro pasticcio. A quando il *mea culpa*? A quando una presa di coscienza seria e dignitosa dello scempio che si sta perpetrando ai danni dell'economia del Paese? Credete, signori della maggioranza, che sia sufficiente una blanda constatazione del vice *premier* Rutelli, sulla necessità di dare ascolto alle preoccupazioni delle categorie vessate da Visco, per riconquistare un rapporto tra fisco e contribuente, volta della lotta all'evasione fiscale? La fiducia del contribuente è fondamentale, per recuperarne anche il contributo. Una lotta che per voi, sino ad ora, ha significato solo burocratizzazione perversa di ogni minimo aspetto della vita economica e lavorativa del cittadino e creazione dell'immagine di uno Stato pervasivo e onnipresente. La lotta all'elusione e all'evasione fiscale non passa per il martirio del contribuente, disincentivato ad adempiere ai suoi doveri di buon cittadino, - al contrario - incentivato a nascondersi per tutelare i propri interessi e ad evadere per poter semplificare. Soprattutto, non possiamo dimenticare che, accanto agli evasori «classici», cioé coloro che volontariamente non dichiarano l'effettivo reddito conseguito, vi è anche chi non lo è per sua volontà, chi rientra nelle ipotesi di evasione interpretativa, generata dal continuo, disorganico e contraddittorio affluvio di norme fiscali, scritte in modo indecifrabile anche per gli esperti del settore e, cosa ancora più grave, con effetti retroattivi,

non per sua volontà, non può rispettare generici ed immotivati redditi predeterminati dall'amministrazione finanziaria, con parametri, coefficienti presuntivi e studi di settore che, ancora oggi, sono male utilizzati dagli uffici, che non rispettano le tassative condizioni di legge che inquadrano questo istituto giuridico come una preselezione alla fase successiva dell'accertamento; una presunzione semplice, che non comporta di per sé stessa alcuna inversione dell'onere della prova a della prova a danno dei contribuenti, che, invece, nella realtà dei fatti, stanno vivendo gravi disagi che li portano giustamente a protestare. La loro protesta sentiamo di dover accogliere.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il Gruppo Per le Autonomie si dichiara soddisfatto per il testo della mozione di maggioranza sulla politica fiscale, in particolare su questo aspetto degli studi di settore; una soddisfazione che nasce anche dal fatto che - mi sia consentito di sottolineare - come Gruppo abbiamo fortemente contribuito alla redazione del testo. Ringrazio in questo contesto le senatrici Thaler Ausserhofer e Rubinato, il senatore Pinzger e gli altri colleghi del Gruppo qui presenti che in prima persona hanno contribuito ad esprimere politicamente una sofferenza sentita dai piccoli e medi imprenditori.

Penso, ad esempio, all'aumento delle pensioni minime e alle politiche di sostegno a favore dei giovani, tutte tematiche non più rinviabili e che come Gruppo per le autonomie avevamo segnalato più volte all'attenzione del Governo. Con la stessa fermezza con la quale abbiamo chiesto e chiediamo l'attenzione ai problemi delle piccole e medie imprese, torniamo infatti a chiedere all'Esecutivo di porre in essere in tempi brevi misure a favore delle famiglie per l'acquisto della prima casa e per la promozione della maternità e paternità. In questo frangente mi sembra doveroso ricordare che le misure che metterà in atto il Governo e quelle che auspichiamo vengano realizzate sono rese possibili grazie all'opera di risanamento dei conti pubblici rigorosamente attuata fin dall'inizio della presente legislatura. Con questa Con questa linea d'azione il Governo non è che abbia guadagnato consenso, il contrario purtroppo, lo si deve dire. L'Esecutivo aveva ereditato un debito pubblico di 1.570 miliardi dai Governi precedenti

Tornando al dibattito sugli studi di settore, riteniamo sia stata fatta la necessaria chiarezza richiesta con forza dalle piccole e medie imprese. Mi consenta, signor Presidente, di aprire una piccola parentesi necessaria per sgomberare il campo da qualsiasi equivoco su polemiche delle scorse settimane. Contrariamente a quanto è stato detto in quest'Aula e scritto sui giornali, il Gruppo Per le Autonomie non si è mai fatto carico di essere interprete di interessi localistici di una o di un altra Regione, come del Trentino‑Alto Adige-Südtirol, come il il collega Eufemi aveva ritenuto; il malessere del mondo imprenditoriale proviene non solo dalle Regioni del Nord, ma ritengo sia un malessere di tutto il Paese intero, sarebbe strumentale - come sanno i colleghi - volerlo circoscrivere solo al Trentino-Alto Adige-Südtirol. Tornando alla mozione dell'Unione, è anche grazie al nostro contributo che si richiede al Governo una revisione degli studi di settore tramite il metodo della concertazione con le categorie interessate. Infatti, i nuovi indici di normalità economica dovranno essere solo sperimentali e non potranno essere usati per accertamenti fiscali automatici. È implicito per noi che nei controlli rimanga, pertanto, l'onere della prova a carico dell'Amministrazione delle finanze e non del contribuente, che deve dimostrare di essere innocente. e questo dovuto confronto tra Governo e categorie, a nostro avviso, si inquadra nella più complessiva cornice da realizzare e nel rispetto scrupoloso dello Statuto del contribuente, creando un nuovo rapporto che non deve prevedere in alcun modo norme retroattive tra il fisco e i contribuenti: questo è uno dei princìpi sacrosanti dello Statuto del contribuente spesso richiamato e richiamato Ma noi ci spingiamo più avanti, traendo esempi da altri Paesi europei, immaginando un fisco non solo ed esclusivamente sanzionatorio: un fisco che accompagni, con un sistema di consulenze, le imprese, al fine di creare un rapporto di fiducia per una nuova, più corretta cultura contributiva. Naturalmente tutto ciò, non esclude in alcun modo le sanzioni, che dovrebbero scattare qualora le imprese, dopo questo percorso consultivo, si dovessero dimostrare recidive. Allo stesso modo, a nome del Gruppo mi preme fugare ogni dubbio riguardo al fatto che la necessaria revisione degli studi di settore non debba assolutamente significare un abbassamento della guardia nei confronti dell'evasione fiscale: questo deve essere e rimane il tema,

vede il fisco impegnato ed è un punto centrale del Governo, in quanto riteniamo che si debba pagare tutti, in modo che tutti possano pagare meno. A tal proposito, siamo soddisfatti che la necessità di abbassare la pressione fiscale anche con i proventi derivanti dalla lotta all'evasione sia stata inserita al primo punto della mozione di maggioranza ed è anche per questo motivo che esprimiamo fin d'ora il nostro voto favorevole a tale mozione. Presidente, ritengo che l'opposizione abbia fatto bene a porre alla nostra attenzione questo tema. Al di là del dibattito, si è riusciti a interloquire e a portare elementi positivi nel confronto e credo che, comunque, lasciamo nei resoconti parlamentari un dibattito importante e ricco. Devo dire subito che siamo per l'applicazione più rigorosa di tutte le misure per contrastare l'evasione fiscale. La situazione che è sotto i nostri occhi, evidenziata in questi ultimi giorni è più disastrosa di quel che si potesse immaginare: oltre la metà delle imprese non è in regola con gli studi di settore. Si è detto che probabilmente è troppo alta la soglia fissata. Personalmente, ritengo che questo sia improbabile, perché oltre la metà denuncia un reddito di impresa di 10.500 euro, cioè 875 euro al mese. È chiaro che qualcosa non funziona. Vi sono comportamenti anomali: magazzini magazzini strapieni, ovviamente magazzini finti o inesistenti, acquisti di attrezzature e macchinari inesistenti, acquisti di materie prime strabordanti rispetto alle vendite dichiarate. Tutto ciò è chiaro che nasconde un'evasione capillare e di massa; tutto ciò costringe i contribuenti onesti (e vorrei che venisse riportata nel resoconto l'affermazione del senatore Galli,

io, Presidente, se vuole) a pagare più tasse del dovuto per tappare i buchi di chi non paga. Se non ci fosse l'evasione fiscale, la pressione fiscale sarebbe più bassa di dieci punti. Gli studi di settore, concordati con le categorie, servono non per chiedere più soldi a tutti i costi, ma per correggere le patologie evidenti ed anomale che ho indicato prima. Chi è in regola non deve temere nulla, chi è sotto la soglia non è obbligato ad aderire. E allora perché c'è stata questa opposizione così ampia, così radicale? Certamente ci sono motivi di convenienza (questo è inutile negarlo), c'è gente che assolutamente non si riconosce negli studi di settore e magari non vuole neanche pagare le tasse, però molti dicono - e credo che questa sia

allora che non sia un problema di scarsa comunicazione, o di comunicazione inefficace: quando la gente e gli operatori in modo così ampio fanno queste affermazioni credo che ci sia qualcosa che non funzioni e quello che non funziona credo sia il fatto che quelli che già pagano le tasse si sentono ulteriormente vessati da più burocrazia e da più adempimenti. A me pare che la nostra mozione chieda sostanzialmente poche cose: prima di tutto la proroga delle scadenze degli studi; prevedere la sperimentalità degli indici di normalità economica; che le anomalie debbano essere approfondite senza accertamenti

realmente la concertazione per individuare le soluzioni tecniche, ma c'è una questione rilevantissima: siamo d'accordo con la concertazione con le parti sociali vedere come è possibile garantire lo stesso gettito, perché qui ci sono 2 miliardi e 700 milioni che ballano e quindi c'è la necessità di avere indicazioni precise al riguardo. Concludo, Presidente, con la questione di ordine più generale. L'opposizione dice che l'unico modo per far pagare le tasse è la riduzione delle aliquote e quindi ridurre la spesa pubblica. Noi diciamo che si può fare, diciamo di sì, se tutti pagano le tasse, perché prima di tutto noi abbiamo un debito, tra l'altro causato ai tempi della Prima Repubblica, e oggi quelli che ci dicono che bisogna ridurre le aliquote e la spesa pubblica sono gli stessi che in quegli anni hanno causato il debito che grava sui conti pubblici del nostro Paese. Dobbiamo garantire servizi essenziali e tutele sociali che sono finanziati dalle tasse, noi siamo per rendere più efficiente la pubblica amministrazione, e quindi ridurre la spesa pubblica partendo dal concetto che la pubblica amministrazione fornisce servizi ai cittadini e i cittadini devono poter essere garantiti e la pubblica amministrazione deve rispondere ai cittadini, non ai partiti che hanno messo quelle persone a lavorare nella pubblica amministrazione. Quindi, più efficienza, più efficacia, più trasparenza, più professionalità. Infine, Presidente, questa è la nostra scommessa: basta con i condoni per fare cassa.

Signor Presidente, colleghi senatori, le mozioni sugli studi di settore mettono in luce le distorsioni create dalla politica fiscale del Governo e della maggioranza di Governo. Cito entrambi questi soggetti di azione politica (Governo e maggioranza parlamentare) perché le lacrime di coccodrillo che diversi esponenti del centro-sinistra stanno versando poco servono a lenire la situazione cui hanno voluto condurre le imprese e le attività produttive italiane. La responsabilità degli atti e delle leggi approvate non può essere sminuita da enunciazioni di principio, ma solo da determinazioni concrete ed efficaci. Una volta in più sono stati contraddetti gli impegni elettorali: con la stessa faciloneria con cui, dismesse le bandiere della pace, la politica estera e militare del Paese ha continuato nella medesima direzione della precedente legislatura, oggi il centro-sinistra ha incrementato la pressione fiscale dopo aver solennemente dichiarato di non volerlo fare. Lo scopo, evidente oggi con la battaglia sulle spoglie del "tesoretto", è quello di consentire di incrementare la spesa pubblica corrente. Così il debito pubblico continua a crescere, né più né meno dell'evasione che con altrettanta e bugiarda enfasi era stato promesso di combattere. Un anno è stato sufficiente per dimostrare quanto vuoti fossero i progetti e i proclami di risanamento della finanza pubblica e di crescita e sviluppo che ci erano stati ammanniti pochi mesi orsono, tanto che oggi i numeri ci mettono fanalino di coda dei Paesi dell'Unione Europea. Questo è stato, in maniera particolarmente efficace, denunciato dai presidenti di Confartigianato e Confcommercio durante le ultime assemblee generali. Ma eccoli i numeri che ci interessano, i numeri della verità. entrate fiscali sono in aumento di 6,7 miliardi tra i primi quattro mesi dell'anno in corso rispetto all'identico periodo dell'anno precedente; l'incremento su base annua tra 2006 e 2005 si è attestato sul 7,7 pressione fiscale supera la media europea, poco invidiabile primato, che ci porta dal 40,6 al 42,3 per cento. Naturalmente queste sono le cifre che riguardano la pressione fiscale "apparente", "apparente", perché quella "reale", cioè quella sui soli redditi dei contribuenti onesti, supera il 50

debito pubblico a marzo 2007 supera di molto la soglia dei 1.600 miliardi, con un incremento di 43 miliardi rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'evasione è stabile a 270 miliardi l'anno, secondo i dati dell'ufficio studi dell'Agenzia delle entrate, o più. Secondo la CGIA di Mestre in Italia nel 2006 si stimano 311 miliardi di evasione: 200 nel lavoro sommerso, 100 nell'economia criminale, 7 nella grande impresa, 4 nel lavoro autonomo e nelle professioni. Anche se non si dispone di proiezioni per l'anno 2006, i dati forniti dalla Guardia di finanza nella lotta contro l'evasione ci permettono di comprendere la realtà dei fatti.

nel 2006 a 16.883 milioni di euro. Evasori totali e paratotali scoperti nei rispettivi anni: 8.421 nel 2005, 7.288 colleghi senatori, è la sconfitta nella lotta all'evasione la prova che il maggior introito fiscale proviene dall'aumento della pressione e rimane a carico di chi ha sempre pagato! Questi sono i numeri, impietosi, di un doppio fallimento: da un lato quello della gestione delle entrate e della spesa pubblica, dall'altro quello della lotta all'evasione. Al centro del campo di tiro, un vero e proprio poligono, è stata messa la piccola impresa, l'impresa artigianale, il commercio al minuto, il lavoro autonomo, il professionista, cioè l'asse portante dell'economia di questo Paese. la verità è che gli indicatori elaborati dal vice ministro Visco deformano la realtà in maniera totalmente arbitraria. Secondo l'ufficio studi dell'Agenzia delle entrate, nella dichiarazione dei redditi 2005, cioè

Sono vergognose ed offensive le illazioni del vice ministro Visco e anche quelle che ho sentito poco fa del collega Ripamonti, che hanno tentato di additare all'opinione pubblica il mondo della libera imprenditoria e della professione come fonte

Non basta certo il pannicello caldo della mozione che il centro-sinistra vuole approvare questa sera, che è una vera e propria presa in giro. Questa mozione infatti non toglie nulla all'efficacia concreta della politica fiscale vessatoria del Governo sin qui attuata; anzi, con il proprio disposto ne avvalora ulteriormente finalità e metodi. Le risposte concrete che corrispondono alle attese di contribuenti onesti si trovano chiare e indelebili nella mozione presentata dalla Casa delle Libertà e in quella di Solo in queste mozioni si impegna il Governo ad eliminare ogni effetto retroattivo sui redditi del 2006 dei nuovi indicatori di normalità e degli studi di settore e ad aprire il tavolo negoziale con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, con lo scopo di concordarne la revisione. Votando queste mozioni, si darà al Paese un messaggio chiaro e inequivocabile, nei confronti del quale ognuno deve assumersi la propria responsabilità. La Lega Nord sarà dalla parte della gente che lavora e che produce, e naturalmente dalla parte della Padania.

il Gruppo della Sinistra democratica per il socialismo europeo ha sottoscritto la mozione della maggioranza e la sostiene in modo convinto. Il senatore Galardi, nel suo intervento in discussione generale, ha esposto la nostra posizione in modo articolato. Ad essa faccio riferimento, limitandomi ad alcune considerazioni sommarie. Noi riteniamo indispensabile proseguire la lotta all'evasione e all'elusione fiscale e al tempo stesso avvertiamo l'esigenza che queste politiche di rigore siano contemperate con un senso di giustizia e con la ricerca di un nuovo rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. I dati recentemente resi pubblici sull'entità dell'evasione e sul modo inaccettabile con cui sono oberati oltre il dovuto i contribuenti onesti rendono necessario un impegno su entrambi i fronti, sotto entrambi gli aspetti. Dico molto chiaramente noi rifiutiamo la rappresentazione del Paese che punta ad una contrapposizione fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi; respingiamo come scandalosa la taccia di fannulloni che è stata rivolta ai lavoratori dipendenti: vadano a dirlo a quei lavoratori di Napoli che tutte le settimane devono prendere il treno per andare a lavorare a Milano, e che ieri sono stati costretti a ricorrere a quella certamente non condivisibile forma di protesta. protesta. Al tempo stesso, respingiamo di etichettare come evasori intere categorie di lavoratori, come quelle che operano nel campo del lavoro autonomo: anche questo è lavoro, è lavoro, di cui parla la nostra Costituzione, che all'articolo 1 afferma che «l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». Il lavoro dell'artigiano, il lavoro del piccolo esercente, il lavoro del piccolo imprenditore, il lavoro del professionista merita rispetto, attenzione e tutela. Per questo è necessario che gli studi di settore si qualifichino come uno strumento per la conoscenza sempre più adeguata delle trasformazioni dell'economia italiana e non come una forma surrettizia di reintroduzione della *minimum tax*. tax*. Chiediamo che il metodo del confronto e della concertazione tenga conto di questo mondo del lavoro autonomo. La rappresentanza prioritaria del mondo delle imprese affidata a Confindustria non rappresenta la realtà delle imprese italiane. Già molto e troppo hanno avuto Confindustria e la grande impresa: dal cuneo fiscale, allo stesso impianto di una legge fiscale come l'IRAP che privilegia la grande impresa a bassa densità di lavoro. Ora bisogna tornare allo spirito e alla lettera del protocollo firmato nel dicembre scorso, il quale prevede che gli indicatori di normalità economica siano individuati con la partecipazione degli esperti delle categorie interessate e bisogna che vengano uniformati al protocollo anche gli indicatori di normalità economica individuati con il decreto ministeriale del 20 marzo 2007. Chiediamo, inoltre, al Governo di assicurare certezza del diritto e semplificazioni burocratiche a questi operatori: non si possono spostare termini e dare direttive con comunicati a mezzo stampa, perché in questo modo si creano intralci e difficoltà nel lavoro e nel tessuto della piccola impresa, dell'artigianato, del piccolo commercio che è un tessuto portante della economia italiana. D'altra parte, solo nell'ambito di una sforzo generalizzato e condiviso di lotta all'evasione - e per questo è interesse di tali categorie collaborare - sarà poi perseguibile e giustificabile la diminuzione del carico fiscale e degli adempimenti richiesta dalle famiglie e dalle imprese di coloro che davvero usano usano l'impresa per lavorare. La riduzione del carico fiscale non è un obiettivo da perseguire in modo squilibrato fra ricchi e poveri, fra grandi e piccole imprese: le grandi imprese si sono già giovate di misure *ad hoc*, come il cuneo fiscale che adesso, pare, debba essere esteso persino alle banche e alle assicurazioni. È ora giusto prestare attenzione ai settori più deboli, anche se sempre pretendendo comportamenti improntati a fedeltà fiscale e al rispetto delle leggi. Il nostro voto favorevole alla mozione della maggioranza si accompagna all'invito al Governo ad informare sempre più le proprie politiche economiche e sociali a quel senso di rigore e di giustizia che è indispensabile per rinsaldare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella volontà di cambiamento di cui il centro-sinistra è espressione; una volontà di cambiamento che punta non a dividere il Paese, ma a tenere conto del contributo di tutti alla crescita, allo sviluppo, alla possibilità di un rinnovamento dell'Italia. E dal mondo dell'impresa minore, dell'artigianato, del lavoro autonomo, delle attività professionali, da questo mondo può e deve venire un importante contributo a quest'azione di cambiamento.

l'argomento oggi in discussione è di fondamentale importanza per gran parte del mondo produttivo del nostro Paese, perché riguarda il lavoro autonomo e le piccole e medie imprese; e credo che ad oggi nessuno possa negare la gravita della situazione che si è determinata a seguito della gestione maldestra da parte del Governo degli studi di settore. Ancora una volta la politica fiscale è stata usata come una mannaia che si è abbattuta indiscriminatamente su tutti i contribuenti rischiando di mettere in ginocchio tanti lavoratori onesti e tante piccole aziende (pensiamo, in particolar modo, ai contoterzisti) che, con enormi difficoltà, sono riuscite ad andare avanti superando i mutamenti strutturali dovuti alla globalizzazione. Ma sembra che questo Governo, piuttosto che sostenere e incentivare una ripresa economica che non si è ancora consolidata, continui a mettere in atto politiche punitive e vessatorie! La vicenda degli studi di settore è emblematica dell'incapacità di governare di questo Governo e della sua maggioranza: tutto ciò che di sbagliato si poteva fare è stato fatto. Vi è stata un'*escalation* di errori che alla fine ha esasperato le categorie coinvolte e che ha generato un coro di proteste unanime. È stata sbagliata la scelta di inserire in finanziaria i nuovi indici di normalità prevedendone l'applicazione, peraltro retroattiva, al periodo di imposta precedente, come è stata sbagliata la scelta di adottare questi indici unilateralmente, senza alcun confronto con le categorie di professionisti del settore, contravvenendo, caro senatore Salvi, all'accordo raggiunto nello scorso mese di dicembre di avviare un dibattito sulla revisione degli studi. Sia nel merito che nelle modalità la questione è stata trattata nel modo peggiore, generando solo confusione e malcontento generale. I nuovi indici di normalità retroattivi, definiti in modo astratto, hanno fatto schizzare i ricavi medi talmente verso l'alto che ben più della metà delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi non risultano a tutt'oggi congrui. E ciò costituisce la prova lampante che qualcosa non ha funzionato e che il sistema non è affidabile perché non corrisponde alla realtà. Di fronte a questo era inevitabile la protesta e la denuncia fatta sia dai contribuenti che dai professionisti addetti alle dichiarazioni dei redditi. E noi abbiamo appoggiato e sostenuto questa protesta non certo per demagogia, ma perché siamo dalla parte dei tanti contribuenti onesti, che sono i più colpiti da questa situazione e che si trovano in enorme difficoltà di fronte a delle regole che vengono cambiate in corso d'opera, nel giro di breve tempo, e senza alcun confronto. Se l'intento era quello di combattere l'evasione, il risultato è stato paradossale perché le vere vittime sono proprio i contribuenti che pagano. Viene il sospetto che l'unico obiettivo di questo Governo è quello di fare cassa a tutti i costi e con qualsiasi strumento possibile, colpendo indistintamente tutti. Gli studi di settore sono stati, quindi, del tutto snaturati e hanno perso la loro iniziale funzione di strumento voluto fortemente anche dalle associazioni di categoria delle imprese per rendere il fisco più equo, fornendo indicatori obiettivi ai contribuenti, e hanno man mano assunto la funzione di idrovora fiscale. La retroattività degli indici di normalità economica, la loro definizione unilaterale stanno chiaramente a testimoniare il fatto che l'unico obiettivo era quello di aumentare il gettito e non certo quello di perfezionare gli studi di settore. E non basta che il vice ministro Visco, di fronte alla confusione creatasi e alle legittime proteste, si sia affrettato ad affermare che non si tratta di una *minimum tax* perché non sussiste l'obbligo di adeguarsi ai risultati degli studi: sappiamo bene che in sede di accertamento, che scatta automaticamente, è difficile per il contribuente giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli previsti. Per cui non resta che pagare la differenza o andare incontro al contenzioso con tutto quello che ciò comporta in termini di costi, di tempo, e di incertezza del risultato. E non sono neanche sufficienti ad uscire dall'*impasse* i rimedi proposti in questi giorni - e che sono previsti anche dalla mozione della maggioranza - tesi a considerare sperimentali gli indici o a sterilizzarli: si tratta di palliativi che non servono a ricondurre la questione alla normalità e alla ragionevolezza, come è invece sarebbe ed è necessario. Occorre azzerare - ripeto - azzerare la situazione e ripartire da capo. Occorre cioè sospendere l'applicazione degli indici di normalità, come richiesto a gran voce dalle categorie interessate, e applicare per il periodo d'imposta del 2006 gli indici di congruità come stabiliti in precedenza. Successivamente è necessario avviare un'ampia revisione degli studi di settore che, se utilizzati nella giusta direzione e con gli opportuni correttivi, possono davvero costituire uno strumento valido ed efficace per instaurare un rapporto equo tra fisco e contribuente. Ma affinché ciò avvenga è necessario agire ed aprire un tavolo di confronto con le categorie interessate, che conduca a decisioni condivise e, soprattutto, a criteri e indici che riflettano le reali condizioni delle varie categorie produttive e che, quindi, mettano tutti nelle condizioni di pagare quanto equamente equamente dovuto. La lotta all'evasione fiscale, infatti, è un obiettivo prioritario per tutti, ma deve essere perseguito con gli strumenti idonei e andando a colpire le vere sacche di evasione; non si può certo pensare di vessare tutti indistintamente, cambiando i criteri di riferimento fiscale fissati per ogni attività in modo retroattivo. La correttezza del rapporto fisco-contribuente non può essere a senso unico, ma deve valere anche e soprattutto per lo Stato. Questo è secondo noi l'unica strada da seguire per tutelare quei lavoratori autonomi e quelle piccole e medie imprese che, rimanendo così le cose, si troverebbero in enormi difficoltà, essendo costrette a pagare somme abnormi, che non rispecchiano assolutamente la realtà economica del Paese e che avrebbero conseguenze negative sull'intero sistema economico. E per questo l'UDC voterà con convinzione a favore della mozione a prima firma Schifani, D'Onofrio ed altri, che va proprio nella direzione di porre un rimedio efficace agli errori commessi: azzerare quindi, sospendere, aprire un tavolo di confronto con le categorie! Questo significa governare; il resto è solo squallida improvvisazione!

abbiamo risposto a una sollecitazione che ci viene dalle categorie direttamente interessate, quanto per il fatto che richiama all'attenzione di noi tutti la presenza di una questione fiscale, che non è questione ragionieristica e astratta, ma è sostanzialmente il mezzo attraverso cui una società organizza gli strumenti della propria coesione sociale. È evidente che tutte le posizioni che mirano in maniera esplicita a considerare il prelievo fiscale una vessazione, un'assurda pretesa dello Stato, una forma di arbitraria intromissione nella libertà dei singoli di intraprendere e di guadagnare pensano in fondo a una società in cui, come nella legge della giungla, il più forte sopravvive e il debole, non avendo strumenti e risorse, soccombe. Questo è il punto, e tale aspetto, considerato un elemento di modernità da parte di chi lo sostiene, in realtà rappresenta un elemento di forte debolezza. di forte debolezza. Proprio per questo, dobbiamo essere in grado di riaffermare il principio che il fisco, come dice la Costituzione, va pagato da tutti coloro che possono e deve consistere

orientato a rispondere a quel criterio di progressività e proporzionalità di cui parla la Costituzione. È evidente che questo strumento, che per cinque anni è rimasto negletto e senza manutenzione, nel momento in cui con la finanziaria del dicembre scorso è stato implementato con

delle pecche serie che vanno corrette. In questa direzione va la mozione che abbiamo presentato, di cui anche io sono firmatario, sostanzialmente rivolta ad

firmato un protocollo d'intesa con le associazioni, proprio per definire le modalità di applicazione di questi strumenti più raffinati quali sono gli indicatori di normalità economica.

abbia creato malessere, sconcerto perché tutti gli interventi che hanno una dimensione media ovviamente possono essere, e sono, inadeguati per eccesso per una gran parte di contribuenti, e per difetto per una parte, magari piccola, di contribuenti. Mi metto nei panni di quegli artigiani, di quei piccoli imprenditori, di quei commercianti che sono stati fedeli all'obbligo fiscale, e mi rendo conto che giustamente, di fronte ad un incremento che li mette in condizione di difficoltà, protestino.

della necessità di correggere ciò che non va, mi rendo conto che non siamo in presenza di un atto generalizzato di vessazione ma di interventi che hanno bisogno di una correzione. Non dimentichiamoci, peraltro, che a fronte di 4 milioni di lavoratori autonomi, soggetti agli studi di settore, ci sono oltre 20 milioni di lavoratori dipendenti

Signor Presidente, mi consenta di esprimere la mia personale solidarietà al sottosegretario Lettieri: gliel'ho detto prima privatamente e ora la esprimo qui in pubblico. Mi evoca molto l'immagine, con tutte le differenze storiche del caso, di quando Alcide De Gasperi andò alla Conferenza di Parigi e fu costretto a dire che si rendeva conto che tutto, salvo la personale cortesia Qualche giorno fa, il Presidente del Consiglio ha detto che in Italia c'è un'aria irrespirabile. Credo che il Presidente del Consiglio abbia ragione. Ho illustrato nella discussione generale in precedenza le ragioni macroeconomiche con le quali il suo Governo ha reso l'aria irrespirabile in questo Paese, truccando i conti e procedendo, ancora questa sera, con un bilancio falso dello Stato e con falsi numeri di finanza pubblica. Vorrei ora aggiungere però alcuni elementi microeconomici, perché forse ci siamo abituati in fretta (ha diffuso un gas soporifero che sembra addormentare la sua stessa maggioranza) ma molti dei problemi che abbiamo discusso in quest'Aula derivano semplicemente dal fatto che il Governo prende decisioni cervellotiche e demenziali senza neanche rendere consapevole la sua stessa maggioranza, consapevole la sua stessa maggioranza, che spesso deve correre ai ripari cercando di convincere il Governo a mettere qualche pezza. Faccio pochissimi esempi: i *ticket* nel settore della sanità. Siamo arrivati ad annunciare sulla stampa che il Governo Prodi l'aveva eliminato, senza dire che il Governo Prodi l'aveva introdotto qualche giorno prima. E siamo da capo con gli studi di settore; questo provvedimento retroattivo, in particolare per l'anno 2006, causa quella ipocrisia gigantesca di cui ho già riferito nel precedente intervento. Tuttavia, amico sottosegretario Lettieri, dire che non scatta automaticamente l'accertamento significa commettere un'altra ipocrisia perché certamente l'accertamento non ci sarà se il contribuente si adegua agli indici di normalità; il che vuol dire che automaticamente permane il *vulnus* dell'inversione dell'onere della prova, perché se io mi adeguo, soggiacendo al sopruso e alla vessazione di questi indici retroattivi, non ho l'accertamento, mi metto al riparo ancora una volta. Ciò vuol dire che chi non si adegua vede aumentare enormemente la probabilità dell'accertamento, anche se non scatta automaticamente. Il punto chiave è che occorre eliminare questa retroattività al di là delle ipocrisie della mozione presentata dalla maggioranza che parla di introduzione sperimentale, senza capire qual è la conseguenza operativa di questo, cioè resta la retroattività, il fatto che chi non si adegua deve dimostrare, lui, di avere un reddito non coerente con gli indici di cosiddetta normalità. Un'ipocrisia contenuta ulteriormente nella mozione della maggioranza perché, francamente, cari colleghi della maggioranza, come si fa a scrivere che s'invita il Governo ad abbassare la pressione fiscale, quando il Governo da pochi mesi ha aumentato la pressione fiscale di due punti percentuali e i numeri del Governo dimostrano che non ve ne era affatto bisogno per risanare la finanza pubblica, ma che, forse, oggi ce n'è bisogno perché nel frattempo è esplosa la spesa pubblica corrente a causa delle decisioni di questo Governo e di questa maggioranza? Vengo all'esempio del collega Ripamonti, sbandierato in modo palesemente strumentale dal Governo in questi giorni e, cioè, molti di questi lavoratori autonomi, molti delle Srl dichiarano un reddito di 10.000-11.000 euro l'anno, dichiarano magazzini incoerenti con il fatturato, eccetera. Ammesso che questo sia vero, e non tutto è vero dal lato del prelievo fiscale, collega Ripamonti, le segnalo due elementi sul fronte della spesa pubblica che meriterebbero quantomeno la stessa attenzione con la quale vi dedicate al fronte delle entrate fiscali. Voi avete deliberato in finanziaria un aumento da 107 miliardi a 140 miliardi della voce spesa per acquisti di beni e servizi, 33 miliardi di maggiore spesa pubblica per gli acquisti, dimenticando forse che ci sono parametri simili a quelli citati dal collega Ripamonti sul fronte delle entrate, anche sul fronte della spesa. Quella spesa nasconde 850 euro al giorno di ricovero ospedaliero pagato da ogni contribuente italiano; nasconde 11 siringhe consumate al giorno per ogni italiano ricoverato nell'ospedale pubblico e 38 pillole al giorno, ingerite dal normale degente degli ospedali pubblici italiani. Quella spesa nasconde anche altri 30 miliardi di trasferimenti in conto corrente e in conto capitale alle cosiddette imprese che, in realtà, per il 70 per cento sono le tante IRI locali; avete triplicato il numero delle società, quintuplicato il numero dei consiglieri di amministrazione in queste società. E, allora, la lotta all'evasione è sacrosanta, ma, quantomeno, è altrettanto sacrosanta la lotta alla correzione della spesa pubblica corrente che significa dilapidare le tasse dei contribuenti onesti. Concludo con un'immagine, una vecchia immagine del senatore Andreotti che diceva che quando un orologio è fermo e rotto, almeno due volte al giorno dà l'ora esatta. Mi sembra la rappresentazione di questo Governo: è un orologio rotto che forse due volte al giorno dà l'ora esatta, ma per le restanti 23 ore, 59 minuti e 59 secondi dà l'ora sbagliata all'intero Paese. È per questo che il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore della mozione n.

l'ultima innovazione, prima legislativa con l'articolo 1, comma 14, dell'ultima finanziaria, poi con i decreti ministeriali del 20 marzo, con i quali si sono introdotti questi nuovi «indicatori di normalità economica», si arricchisce ulteriormente il quadro generale di politica fiscale disegnato e, purtroppo, concretamente eseguito da questo Governo. quadro generale di politica fiscale si caratterizza per alcuni elementi fondamentali, tutti dannosi per l'economia e per i cittadini: l'incremento del livello di tassazione, l'istituzione di nuovi e pesanti adempimenti vessatori per i contribuenti onesti e in regola e del tutto inidonei a colpire l'evasione, - cosa ancor più grave - l'applicazione ormai normalmente retroattiva delle disposizioni fiscali. Dirò dopo quale grave *vulnus* questa retroattività costituisce per tutti i cittadini e i contribuenti, ma valutiamo come sono stati introdotti questi cosiddetti indicatori di normalità. Innanzitutto essi sono stati determinati unilateralmente dall'amministrazione finanziaria, riproponendosi così una decisiva questione di carattere teorico. Si ritorna infatti alla posizione Si ritorna infatti alla posizione teorica che vede la pretesa fiscale dello Stato, non un patto costituzionale con i cittadini per provvedere ai servizi collettivi, ma una potestà autoritativa esercitata sulla testa e possibilmente anche contro i cittadini. La cultura liberale e noi stessi dobbiamo opporci a tale impostazione per reintrodurre nel nostro ordinamento una fiscalità elaborata con i cittadini, con le imprese e le loro associazioni ed esercitata in un rapporto di lealtà e di reciproche garanzie. Non bisogna però dimenticare gli aspetti concreti di questi indicatori di normalità; essi infatti costituiscono un passo indietro rispetto agli studi di settore, se solo si riflette sulla circostanza che essi fanno riferimento solo a 200 studi di settore e non ai 2.000 modelli d'impresa individuati per l'elaborazione degli stessi studi di settore. dunque una superficialità, una genericità e quindi la possibilità concreta di colpire contribuenti e imprese oneste. Infine, sono due i più gravi rilievi critici che si devono rivolgere agli indicatori di normalità: in primo luogo essi sono retroattivi. Tanti di noi hanno partecipato all'elaborazione e approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente. Si disse che quella dovesse essere una norma cosiddetta rafforzata, a metà tra la norma ordinaria e la norma costituzionale. In verità, questo Governo fa una prassi sistematica della retroattività della norma fiscale, così venendo meno non soltanto alla norma costituzionale, ma anche e soprattutto allo Statuto dei diritti del contribuente, gettando così nell'incertezza assoluta il contribuente e l'impresa. *(Applausi dai Questi indicatori sono organicamente e strutturalmente inseriti negli studi di settore, così producendosi automaticamente gli effetti che il Governo pretende, e cioè maggiori pretese in termini di ricavi, e dunque di imposte - lo ricordo - di vario tipo, perché incidono direttamente sull'IRES, sull' IRPEF, sull'IRAP, sulle addizionali, ma anche sui contributi e sull'imposta sul valore aggiunto. E non solo, ma essendo strutturalmente e direttamente inseriti negli studi di settore, essi rilevano direttamente sugli accertamenti e con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente: questo è il punto di fondo. Perché è notorio che allorquando lo Stato accerta, sulla base degli studi di settore - ed oggi con gli indicatori di normalità inseriti - lo fa sulla base di presunzioni, ribaltando sul contribuente l'onere della prova, così contribuendo di nuovo ad una vera e propria

i liberali, le imprese e tutti i cittadini devono ribellarsi, di fronte ad una situazione ormai sistematica di questo tipo. Ed allora, francamente inutili e contraddittorie appaiono le imbarazzate proposte formulate dalla mozione della maggioranza. La maggioranza si rende conto che le istanze delle opposizioni sono fondate e allora tenta di contenere, con alcuni articoli della proposta di maggioranza, gli effetti peggiori della introduzione degli indicatori di normalità. Ma come si è già detto, questi tentativi sono inutili e contraddittori, perché gli indicatori di normalità sono stati inseriti strutturalmente - per dire, colleghi - nel *software* degli studi di settore e dunque soltanto la mozione che ha come primo firmatario il presidente Schifani può, con la sospensione degli indicatori di normalità ai fini dell'accertamento e con una generale rinegoziazione con i cittadini, le imprese, le associazioni di categoria, garantire che quegli effetti non si producano. Solo quella mozione riveste le caratteristiche necessarie perlomeno per rimediare al grave *vulnus* che ancora una volta viene inferto - lo ribadisco - ai contribuenti onesti e non agli evasori. Per questo dichiariamo il nostro voto a favore della mozione n. 110 e contro

Chiediamo di riaprire subito il tavolo di confronto, ritornando allo spirito e alla lettera dell'accordo sottoscritto il 14 dicembre dal Governo e dalle categorie rappresentative del lavoro indipendente. Quell'accordo prevedeva, tra l'altro, l'aggiornamento degli studi di settore, la definizione comune dell'istituto di normalità economica per individuare le anomalie che caratterizzavano 400.000 lavoratori autonomi su 3,6 milioni: c'era cioè l'intesa di combattere insieme l'evasione. Voglio ricordare che gli studi di settore sono un importante parametro di riferimento per definire il reddito del lavoro autonomo. È una metodologia utile per i contribuenti e per l'amministrazione fiscale. Ha permesso in passato di liquidare strade sbagliate, come erano quelle della *minimum tax* e quella dell'accertamento induttivo. Bisogna sapere, però, che gli studi di settore si basano sulla collaborazione con le categorie interessate, vanno maneggiati con grande cautela. I risultati degli studi di settore sono come le previsioni meteorologiche: possono a volte non coincidere con la realtà. Con l'accordo del 14 dicembre si è proposto di utilizzare gli istituti di normalità economica per accertare in modo trasparente i soggetti che avevano alterato la realtà. È avvenuto che, fatto l'accordo, mentre era in corso tra l'amministrazione e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori autonomi la revisione di 70 studi di settore e mentre si organizzavano seminari comuni tra associazioni e Agenzia delle entrate per dare una organizzazione efficiente all'istituto del contraddittorio, improvvisamente, nel mese di marzo, è stato deciso unilateralmente dall'Agenzia di applicare e di estendere l'istituto di normalità economica in modo anormale a tutti i contribuenti. Non abbiamo condiviso, e già nella Commissione finanze l'Unione ha proposto il differimento dei termini di pagamento e la sperimentalità degli studi di settore e devo dare atto che il Governo ha dato un primo esito positivo a questa risoluzione della maggioranza. Sappiamo però che ciò non è ancora sufficiente: gli istituti di normalità economica non hanno lo stesso livello di approfondimento e di elaborazione

compiuto è che, estendendo automaticamente gli istituti di normalità economica a tutti i soggetti, ci siamo trovati di colpo a trasformare quelli che erano congrui in incongrui e il livello dei non congrui e degli incoerenti è salito dal 29 al 50 cento. Un'altra criticità che abbiamo presente è che nei requisiti di normalità economica è problematico l'utilizzo dell'indice di valore aggiunto per addetto dobbiamo ascoltare le ragioni che vengono sollevate dalle organizzazioni, in particolare da quelle dell'artigianato. Ecco perché ora nella nostra mozione proponiamo che, dopo le modifiche già apportate dal Governo sulla base della risoluzione che prima ricordavo, senza equivoci gli istituti di normalità economica abbiano una natura sperimentale e che perciò non ci sia alcun automatismo accertativo. Questi istituti devono preservare la funzione originaria di segnali di anomalia meritevoli di approfondimento; insomma, insisto, non ci deve essere, non ci può essere nessun automatismo accertativo, non possono essere, perché sperimentali, punti di riferimento per l'accertamento. Ecco perché, mentre apprezzo le proposte della opposizione, che invita a riaprire immediatamente un tavolo di negoziato, non mi convincono le proposte di sospendere, di annullare o di rinviare gli studi di settore. I problemi ci sono, siamo nel pieno delle dichiarazioni dei redditi: i problemi vanno risolti e non rinviati e chiedere di avere immediatamente un tavolo di negoziato significa proprio dare una risposta ai problemi che abbiamo dinanzi. Non Non condivido, e per la verità non sono stati presenti nel dibattito odierno e non rappresentano nemmeno la posizione delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori autonomi, l'idea di buttare via gli studi di settore. Come si potrebbe dire, parafrasando un vecchio detto, non si butterebbe l'acqua sporca insieme al bambino mantenendo l'acqua sporca: si commetterebbe un grave errore perché non realizzeremmo una iniziativa concreta nei confronti della lotta all'evasione fiscale. Vorrei adesso esporre alcune considerazioni di carattere generale. Non vogliamo trascurare una componente essenziale dello sviluppo contemporaneo qual è quella del lavoro indipendente e sappiamo che nella lotta all'evasione fiscale, nella quale si richiede la collaborazione e il coinvolgimento di tutti, non aiuta, e dobbiamo quindi quindi archiviare una volta per tutte la criminalizzazione di intere categorie, perché combattere l'evasione e la frode fiscale, ripeto, è nell'interesse di tutti. Sappiamo che esiste e resiste nel nostro Paese una opinione secondo la quale i lavoratori indipendenti sono reputati secondari, destinati a scomparire sotto l'incalzare della modernità, Non è così: il lavoro autonomo non è un residuo del passato, ma piuttosto un *mix* di vecchio e di nuovo, di categorie protette e di tante, tantissime piccole imprese fortemente innovative e competitive. e competitive. Dobbiamo sostenerle perché è nell'interesse del Paese, in quanto hanno contribuito molto alla ripresa che è in atto. La mozione - e mi avvio alla conclusione - opera anche alcune scelte strategiche: quella di ritornare sulla strada maestra della concertazione, quella di rispettare lo Statuto del contribuente. È vero, è stato troppe volte violato nella passata legislatura... *(Vivaci proteste dai banchi

La violazione dello Statuto del contribuente è stata il frutto avvelenato della politica di emergenza, ora ci sono le condizioni economiche e politiche per rispettarlo e il Governo deve sapere che l'Unione non chiuderà gli occhi e sarà rigorosa paladina della difesa dello Statuto del contribuente. Ancora segnali importanti, mi scusi, signor Presidente,

Metto ai voti la mozione n. 110 (testo 2) del senatore Schifani ed altri, con l'avvertenza che l'eventuale approvazione preclude i punti 3, 4 e 5 del dispositivo della mozione n. 114 della senatrice Finocchiaro ed altri, nonché il punto 2 del dispositivo della mozione n. 117 del senatore Calderoli ed altri, in quanto l'eliminazione di ogni effetto retroattivo sui redditi 2006 dei nuovi indicatori di normalità economica esclude ogni altra soluzione alternativa più affievolita.

Gli ordini del giorno G1 e G2 (testo 2) del senatore Calderoli non sono, invece, né preclusi, né assorbiti dall'approvazione o dalla reiezione della mozione Schifani. Passiamo

Prima di passare alla votazione della mozione n. 114 della senatrice Finocchiaro avverto gli onorevoli colleghi che la sua eventuale approvazione preclude la votazione del punto 2 del dispositivo della mozione n. 117 del senatore Calderoli ed altri, in quanto si individuano soluzioni relative all'applicazione degli indicatori di normalità economica alternative alla loro mera sospensione.

presentata il 19 giugno 2007, che riguarda la volontà di chiudere il centro tumori di Palazzo Baleani, una struttura sanitaria pubblica che dovrebbe passare da centro tumori a ufficio amministrativo. La sollecito, quindi, a far venire il Ministro a rispondere a questa interrogazione.